Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo l'illustrazione, la discussione e le dichiarazioni di voto. Ricordo che su entrambe le mozioni il Governo ha espresso parere favorevole. Prima di passare alle votazioni, avverto che, essendo le mozioni di contenuto sostanzialmente analogo, l'eventuale approvazione della mozione n. 48 non avrebbe effetto preclusivo nei confronti della successiva, mentre l'eventuale reiezione della prima mozione non consentirebbe la votazione della mozione n. 57.

dopo l'intervento del Ministro della giustizia avrà luogo il dibattito, i cui tempi sono stati stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi riunitasi ieri e già resi noti. Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, senatore Mastella.

Signor Presidente, colleghi senatori, nell'esporre ieri alla Camera lo stato dell'amministrazione della giustizia e il progetto che ho in mente per la sua riforma, ho affermato che le iniziative che sto intraprendendo sono tutte volte a riannodare in tempi rapidi il rapporto di fiducia tra giustizia e cittadini. Il baricentro della mia azione di governo è senza equivoci quello di ottenere processi più rapidi,

Il miglioramento dell'assetto complessivo del sistema giudiziario del processo giova all'intero Paese, del quale la giustizia costituisce un fattore essenziale di sicurezza, ma anche di competitività. Proprio per questo ritengo imprescindibile confrontarmi fin da subito con il ruolo centrale del Parlamento e anche con la società civile. Tuttavia, prima di delineare i tratti principali dei progetti di riforma che mi accingo a presentare al Consiglio dei ministri, sento anche di fronte a voi, onorevoli colleghi, la necessità di richiamare e far mio il monito rivolto dal Capo dello Stato nel suo messaggio di fine anno, cioè quello di un dialogo e di un confronto politico sereno.

dicendo che, in linea con il pensiero del Capo dello Stato, ho condiviso l'impegno per energiche iniziative sui tempi della giustizia, espresso da una specifica risoluzione proposta dall'opposizione - questo è avvenuto alla Camera - accettandone dunque la parte dispositiva. Un acuto malessere che si avverte nel Paese non porta soltanto a ricevere un giudizio negativo da parte dei nostri concittadini: su questo il sistema giudiziario è tra quelli verso i quali il livello di fiducia e di affidamento delle persone è sceso negli ultimi anni in modo significativo, anzi più significativo, e continua a produrre nell'opinione pubblica segni di insofferenza, di incomprensione e, a volte, anche di rancore. Ciò che mi preoccupa di più è proprio l'insoddisfazione che i cittadini traggono dal rapporto con il sistema giustizia. Un'ampia sensazione sotto gli occhi di ciascuno di noi è la diffusione di sentimenti di impotenza, se non di vera e propria rabbia, capaci di favorire la progressiva presa di distanza dei cittadini, non solo dalla giustizia, ma più in generale, ahimé, nei confronti dello Stato e delle istituzioni repubblicane. Troppo spesso il recente passato è stato caratterizzato da toni al di sopra delle righe che, anche in materia di giustizia, hanno reso assai difficile il percorso virtuoso indicatoci di recente con tanta autorevolezza dal Capo dello Stato. Per quanto mi riguarda, la centralità del sistema di giustizia, vero pilastro dell'ordinamento democratico per la difesa dei diritti individuali e la sicurezza dei cittadini, la sua straordinaria importanza per la competitività economica del Paese,

attento - credo - esclusivamente al merito dei problemi, delle proposte e delle possibili soluzioni, con la concretezza imposta da una situazione non più tollerabile per nessuno. La giustizia è tema di tale importanza, crocevia istituzionale di tale delicatezza, che la sua riduzione a semplice occasione per marcare una discontinuità con il recente passato contrasta profondamente con la mia cultura, il mio il mio modo di fare politica e di concepire la vita delle istituzioni. Ritengo quindi auspicabile anche in quest'Aula che il percorso dei disegni di legge che il Governo si accinge a presentare (anzi già oggi ho depositato quello che riguarda l'ordinamento giudiziario

dalle parole che mi arrivano in maniera incomprensibile. A questo proposito, darò conto nel mio intervento di alcuni stimoli ulteriori che ho raccolto nella discussione di ieri alla Camera,

Dirò subito, a chi ha paragonato i miei propositi ad una sorta di libro dei sogni, ad una stravagante utopia, privi l'uno e l'altra di riscontro in concrete proposte, che il termine ragionevole cui intendo fare riferimento è la diretta, ragionata conseguenza del complesso di interventi legislativi e organizzativi che costituiscono il cuore del progetto che mi accingo ad illustrarvi. Voglio anche dire con forza che la stella polare della mia azione di governo sono i cittadini, con il loro bisogno di una giustizia rinnovata ed efficace ma pur sempre autonoma e indipendente nell'esercizio di tutte le sue funzioni, nonché responsabile della qualità del servizio offerto al Paese. Verso di loro sento il dovere di un'iniziativa riformatrice che intendo sostenere con coerenza dinanzi al Parlamento e, spero, con la stragrande maggioranza del Parlamento, in adempimento ai compiti affidatimi dall'articolo 110 della Costituzione e nel pieno rispetto del programma con il quale la mia maggioranza si è presentata di fronte agli elettori. Sono convinto che l'insoddisfazione montante, questa sorta di collera costante, tra gli utenti e gli stessi protagonisti nel mondo giudiziario e del mondo giudiziario si possa arginare soltanto con progetti complessivi e coerenti che incidano sugli aspetti problematici del sistema giustizia che pesano di più sulla collettività. I processi hanno bisogno di tempo per concludersi con una decisione giusta, ma è evidente, e purtroppo amaramente sperimentato, che una durata eccessiva indebolisce fortemente la loro capacità di fare giustizia: quando una sentenza arriva dopo tantissimi anni, anche quando essa è giusta, dà l'idea di una giustizia fortemente ingiusta. È una situazione che ha del paradossale: senza la disponibilità di tempo adeguato si rischia la sommarietà di ogni giudizio (e non è questa l'idea con la quale convengo), ma con un tempo eccessivo si ha inevitabilmente la frustrazione dell'aspettativa di giustizia. Al paradosso ci si sottrae forse realizzando e mantenendo in piedi, nella legislazione e nella prassi degli attori processuali, il difficile equilibrio espresso dalla qualificazione costituzionale di ragionevolezza della durata dei processi giusti. I tempi dei processi non possono che essere una priorità della politica e delle categorie professionali che per il processo operano, quindi i magistrati e gli avvocati innanzi tutto, ma, sempre con lo sguardo rivolto ai cittadini, avvocati e magistrati cospirano a rendere certa ed efficace la giustizia rispetto al cittadino come tale. Al riguardo, debbo dire che l'Europa da anni, attraverso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo e lo stesso Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, esercita (ma inutilmente fino ad ora) una forte pressione sul nostro Paese perché si faccia qualcosa e si dia la necessaria effettività al diritto ad un giusto processo. Ma il problema è, se si vuole, più grave. Non si tratta soltanto di dare una risposta alla Comunità Europea perché siamo diventati più europei, perché c'è maggiore cooperazione europea, perché c'è minore allergia rispetto a quello che avviene in sintesi comunitaria: assolutamente no, anche se ritengo che questo sia un dovere politico inderogabile. In gioco vi è qualcosa in più: è in gioco, infatti, a mio parere, la stessa tenuta del sistema democratico del Paese, l'effettività della tutela dei diritti, che ne è condizione imprescindibile, e insieme la credibilità stessa della giustizia nei confronti e agli occhi dei cittadini. Quindi, siamo ai costi, non solo legati all'esborso di danaro necessario per l'accesso alla giustizia, ma anche e forse soprattutto al negativo impatto su individui e società che i ritardi nella resa giustizia producono. Infine, la stessa certezza del diritto, sovente messa in discussione anche in questi giorni dall'intreccio tra mediatizzazione e taluni comportamenti di singoli attori. Fronteggiare, allora, questa crisi di affidabilità della giustizia non è solo una priorità del Governo, che la ritiene sua. Del resto, questa priorità è stata enunciata anche di recente dal Presidente del Consiglio nel conclave, o nella sorta di *meeting*, svoltosi a Caserta.

Nell'esporre sinteticamente quanto nel corso del 2006 si è verificato nell'amministrazione della giustizia (mi trovo a mezz'aria, tra il già e il non ancora, tra quanto hanno compiuto e determinato agli atti di politica giudiziaria il Governo precedente ed il mio, in quanto siamo a metà di questo guado, di questo passaggio giudiziario), giudiziario), per la parte che ha riguardato il mio predecessore e per la parte che riguarda me limiterò il mio discorso ad alcuni nodi ed elementi essenziali. Rinvio, per quanto mi riguarda, al più completo e complesso documento inviato ai Presidenti delle Commissioni giustizia e affari costituzionali e al Presidente del Senato,

Tali dati non sono certo ancora sufficienti, nonostante i ripetuti annunci del precedente Governo, a rispondere all'esigenza di disporre di strumenti di misura e conoscenza idonei a consentire una valutazione esatta delle *performance* complessive e di settore del sistema giudiziario. Dotare l'amministrazione di affidabili strumenti di rilevazione statistica è un campo nel quale impegnare con decisione in futuro l'azione dell'intero Governo. È noto che il Parlamento ha provveduto, su mia proposta, ad adottare un provvedimento di parziale sospensione (e questo ramo del Parlamento ha contribuito a ciò in maniera più efficace dell'altro).

Sono noti i conflitti e le tensioni laceranti che quella riforma aveva prodotto nel tessuto istituzionale, mettendo a rischio, probabilmente, i princìpi fondamentali di autonomia (così era stata censita quella riforma), e indipendenza della magistratura.

è stata quella di riportare serenità, evitando inutili litigiosità istituzionali. L'intervento del Parlamento ha rappresentato, a mio avviso, un atto di grande responsabilità

Passo a dettagliare, come esprime la legge a motivo della quale sono oggi in Senato, i dati riferiti alla giustizia civile per il corso di quest'anno. I dati statistici riferibili al 2005 e al dato tendenziale annuale rilevato al giugno 2006 indicano un costante aumento della domanda di giustizia. Le cause iscritte nel 2005 sono state 4.330.305, a fronte, nel precedente anno, di 4.252.875 cause. La capacità di risposta del sistema a tale aumento reagisce secondo un tasso di incremento pari a circa il 2 per cento annuo, in linea con l'evoluzione registrata nel quinquennio.

Le previsioni per il 2006, sulla base del dato del primo semestre, non si discostano in modo significativo da quanto finora osservato, con un aumento di procedimenti esauriti presso le corti d'appello e i giudici di pace ed un sostanziale equilibrio del dato per tribunali e tribunali per i minorenni. Il dato da sottolineare e che pongo alla vostra attenzione, onorevoli senatori, per comprendere l'ineludibilità e l'assoluta urgenza di scelte deflattive forti è che, nonostante il lieve andamento crescente, il numero dei procedimenti definiti ha però continuato a mantenersi, come nel 2004, al di sotto del numero di nuovi iscritti, con conseguente crescita, purtroppo, del contenzioso arretrato; il numero dei procedimenti pendenti sfiora, dunque, i cinque milioni, in area prossima al numero annuale sia dei procedimenti iscritti sia di quelli definiti. Tali dati vanno interpretati in relazione a quelli relativi alla durata prevedibile dei processi iscritti al 2005 (i cosiddetti tempi di giacenza) e nei quali si registra, con poche eccezioni, un peggioramento da un anno all'altro, che può ormai ritenersi cronico: 30 mesi di giacenza media attesa per un processo di cognizione ordinaria iscritto nel 2005 in primo grado a Roma (ma, addirittura, 52 a Messina) o 44 mesi su scala nazionale per la definizione di un analogo processo in appello. Rappresentano questi, onorevoli senatori, indici di durata indegni di un Paese civile, ai quali non credo possiamo tutti assieme consegnarci e rassegnarci.

la giacenza media in giorni, nelle varie tipologie di ufficio, non registra variazioni di rilievo (ad esempio, da 619 a 622 giorni per il dibattimento collegiale in tribunale). La variazione più alta attiene al dibattimento presso il giudice di pace, la cui giacenza passa da 225 giorni nel 2004 a 285 nel 2005. Notevole, poi, la variabilità tra le giacenze dei singoli uffici, secondo territorialità e dimensione: nel caso delle corti d'appello, ad esempio, si passa da 230-250 giorni per le corti di Palermo e di Potenza ai 1.200 giorni di Ancona e Venezia - ascoltate bene! - a fronte di una media nazionale pari a 622 giorni. Anche nel settore penale gli indici disponibili indicano, dunque, la necessità - io credo - di interventi urgenti per garantire il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

e latitudine dal punto di vista della giurisprudenza e delle accademie a vari orientamenti disciplinari. Da loro e con loro tentiamo di portare avanti, trattare, definire dallo studio e dalla topografia ideale a quella normativa determinando cognizioni che possano essere assunte per le diverse discipline processuali e sostanziali. L'urgenza e la gravità dei problemi innanzi descritti necessitano di un vero e proprio piano straordinario per la giustizia, a cominciare dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, a seguito della sospensione verificatasi e approvata dalla maggioranza e non soltanto dalla maggioranza.

questa è una sorta di *mission* impossibile: è vero che siamo nel 2007, quindi lo 007 vale anche per la *mission* impossibile sul piano e nel mondo della giustizia.

allora, che bisogni anche ragionare così: se il Parlamento ritiene che questa idea (l'accelerazione dei processi, un cambiamento ed una modernizzazione per quanto ci riguarda) trovi un grado

verso la fine di quest'anno, perché tale è la traiettoria parlamentare) a determinare anche che vi sia una forma di apporto calorico in termini di risorse necessarie per affrontare il tema del piano straordinario per la giustizia italiana. Gli interventi che io propongo riguardano, dunque, i seguenti temi questo sarà l'architrave su cui imposteremo questa sorta di pacchetto che definiremo abbastanza presto, iniziando come già ho detto, da oggi, e poi nelle prossime settimane, con un progetto complessivo che sottoporrò alla vostra attenzione e al giudizio parlamentare): ordinamento giudiziario (come già ho detto); processo civile; processo penale; misure di organizzazione e razionalizzazione della macchina giudiziaria; correzione delle cosiddette norme *ad personam*. Dico subito - e sottolineo - che il vecchio sistema ordinamentale e la stessa riforma recata dalla legge n. 150 del 2005 non realizzano un adeguato sistema di valutazione dei magistrati. La professionalità del magistrato non può più essere affermata solo per presunzioni e soltanto in occasione dei passaggi di qualifica troppo distanziati nel tempo. Allo stesso modo, questa procedura un po' bislacca e molto bizantina dei concorsi prevista dalla riforma sospesa dal Parlamento non valorizzava adeguatamente l'attività dei magistrati, basando la progressione su esami e titoli teorici e formali, spesso non conferenti con il concreto esercizio della giurisdizione. Al contrario, la mia riforma - spero, onorevoli colleghi, la vostra riforma - punta ad un magistrato più preparato, perché, credo, reclutato nel modo migliore, scelto negli incarichi successivi, perché migliore per le funzioni da attribuire. In altri termini, la previsione di un continuo controllo sulla professionalità e la scelta per gli incarichi direttivi, fondata fondata soprattutto sulle capacità di organizzazione e di gestione degli uffici. C'è stato una sorta di profeta, un po' disarmato in Italia, che si era applicato sul piano della giurisprudenza, Beria D'Argentine, che è stato il primo che ha evocato e sottolineato questi aspetti e la

Pertanto, e parlo sempre ai magistrati, sarà previsto un sistema di selezione più efficace, in cui per accedere alla magistratura non basterà soltanto la laurea ed un concorso teorico. Si tratterà di un concorso di secondo grado ed un corso-concorso, in cui ad una prima selezione teorica farà seguito un corso ed una selezione finale teorico-pratica. Saranno previsti momenti ravvicinati, ogni quattro anni, di valutazione dell'attività dei magistrati, anche con conseguenze di rilievo economiche e di carriera nel caso, sottolineo, di riscontrata inadeguatezza. L'analisi delle capacità organizzative relative agli incarichi direttivi dovrà essere elemento costante della valutazione periodica, da riprendere ed approfondire in occasione della valutazione specifica richiesta per il conferimento di un incarico direttivo. L'esercizio delle funzioni direttive, poi, sarà caratterizzato da un maggiore controllo di professionalità e di gestione, con limiti di tempo ben definiti: quattro anni, ma rinnovabili soltanto una volta. La carriera resta unica, e so di parlare di una cosa che è eretica per alcuni e che mostra, invece, un giudizio di maggior attenzione e propensione da parte di altri. Alla marcata separazione tra funzioni giudicanti e requirenti sussiste un sistema di distinzione delle funzioni, in cui il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa viene consentito, ma resta legato a due presupposti: la frequenza di un corso di qualificazione professionale ed un giudizio di idoneità specifica, con limiti di incompatibilità a livello distrettuale. La Scuola della magistratura si occuperà soltanto della formazione iniziale e continua dei magistrati, senza alcuna invasione di competenze con il Consiglio superiore della magistratura. Il nuovo assetto ordinamentale dovrà essere accompagnato da una riforma del Consiglio superiore della magistratura, i cui componenti dovrebbero essere - e questo è uno degli elementi all'interno della mia riforma - elevati a 30 e la struttura amministrativa potenziata adeguatamente. Ogni processo, e parlo del processo civile, dovrà pervenire a decisione definitiva entro un termine prestabilito, sulla base della giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo per procedimenti dello stesso tipo. La durata di un processo ordinario di media complessità non dovrà oltrepassare i cinque anni nei tre gradi di giudizio: due anni in primo grado, due anni in appello e un anno in Cassazione. So che è una scommessa,

(accusa e difesa, che sono garantite dalla Costituzione, anche se la Costituzione garantisce a parità di condizioni e non tempi all'infinito o meline all'infinito da parte di questi soggetti)

Sono attribuiti al giudice terzo, responsabile del procedimento, poteri officiosi che consentano il governo del processo. In caso di mancato rispetto del termine massimo di ragionevole durata, il magistrato dovrà tempestivamente informare il dirigente del suo ufficio, che avrà sia il dovere di costante controllo, sia l'obbligo di prendere ogni necessaria iniziativa, di carattere organizzativo o anche disciplinare. La valorizzazione del ruolo conciliativo del giudice nella prima fase del procedimento, accompagnata dalla previsione di sanzioni processuali a carico della parte che abbia, senza giusti motivi, rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla controparte o proposta dal giudice, si muovono pure nel senso della responsabilizzazione di tutte le parti di fronte alla domanda della giustizia, di fronte a quanto accertato e garantito dalla Costituzione. Condivido, come già anticipato, l'invito che mi è giunto ieri dal dibattito di fronte alla Camera dei deputati a compiere ogni sforzo ulteriore per impedire che la motivazione dei provvedimenti giudiziari sia sovrabbondante e costituisca, quindi, essa stessa una causa della lentezza del processo: ritengo quindi che vada ragionevolmente contemplata una più diffusa ammissibilità della motivazione succinta della sentenza. Sarà inoltre alleggerito il peso delle questioni di competenza, che tanto alimentano una sorta di gioco dell'oca in andata e in ritorno successivi, prevedendo un procedimento semplificato in luogo del farraginoso meccanismo del regolamento di competenza. Se si considera che solo nel 2005 sono pervenuti alla Corte di cassazione 2.243 ricorsi per regolamento di competenza una sopravvenienza totale di 29.975 ricorsi, si possono facilmente cogliere i riflessi positivi che, anche sul versante più generale della deflazione dei carichi e dei flussi, tale misura può garantire. Sono poi previsti altri interventi sul processo tesi a ridurne la durata. Tra questi, lo snellimento del sistema delle notifiche, l'aumento della competenza per valore del giudice di pace, la semplificazione del regime delle nullità processuali, attraverso la riduzione delle relative ipotesi e il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli. Inoltre, la modifica degli articoli 181 e 309 del codice di rito, in modo che l'assenza delle parti in udienza determini immediatamente la cancellazione della causa dal ruolo, al fine di ovviare ad una delle cause più frequenti di allungamento dei processi; l'introduzione del procedimento sommario non cautelare, per consentire la definizione della controversia attraverso una procedura semplificata e veloce; la trasformazione dell'appello da gravame devolutivo, che consente una nuova delibazione sulla fondatezza della domanda, a mezzo di impugnazione a motivi chiusi e specifici, come peraltro da tempo auspicato dalla migliore dottrina. In tal modo, oggetto dell'appello diventerebbe la sentenza di primo grado eventualmente viziata, come attualmente accade nel giudizio di Cassazione. La razionalizzazione dei meccanismi di liquidazione delle spese processuali, attualmente strettamente purtroppo correlate alla durata (anche se eccessiva) del processo. Il meccanismo di liquidazione dovrebbe essere sganciato dalla durata del processo e, anzi, dovrebbe prevedere incentivi in caso di minor durata, valorizzando così l'impegno in termini di risultato e la qualità anche professionale, a volte, invece, purtroppo scadente da parte di qualcuno. Sono anche convinto della necessità di una sostanziale riduzione dei termini di sospensione del processo nel periodo feriale, che attualmente decorrono dal 1° agosto al 15 settembre e che, con la riforma,

considerato che, negli ultimi anni, si è assistito, per un verso, ad un vero e proprio fenomeno di erosione del modello del processo civile ordinario a cognizione piena e, per altro verso, al moltiplicarsi dei riti speciali. Sarà mio impegno, invece, affrontare anche sul processo penale il problema dell'efficienza e della durata ragionevole del processo**.** Bisogna infatti evitare - usando una metafora sportiva a me particolarmente cara - che qualcuno possa «far melina» nel gioco processuale, sperando di lucrare una pronuncia sulla prescrizione. Nello stesso tempo vanno responsabilizzate anche in questo ambito magistrati, avvocati, periti e personale amministrativo per garantire che il processo penale abbia un termine massimo ben preciso (e il massimo per me è sempre di cinque anni nei tre gradi di giudizio) e non possa superarlo, fatta eccezione per quei processi di particolare complessità, legati all'accertamento di fatti connessi alla criminalità organizzata o al terrorismo. Intendo proporre per l'approvazione un provvedimento legislativo, già elaborato dai miei uffici, che preveda anche nel settore penale la necessaria ed efficace programmazione dei tempi del processo. Questo intervento, nel rispetto degli *standard* imposti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è volto da un lato a garanzia dei diritti delle parti e, dall'altro, ad assicurare la soddisfazione della legittima pretesa punitiva dello Stato, baluardo della libera convivenza civile. In quest'ottica intendo, inoltre, rivedere il regime delle nullità che non incidano sulle garanzie di difesa. Ho visto che vi è una grande discussione sui tempi e quant'altro, ma voglio rassicurare la classe forense: non viene seguito nessun criterio per il quale si possa penalizzare la difesa come tale, ma ampliare, se possibile, le garanzie di difesa, porle comunque sulla stessa tenuta in maniera rigorosa di quanto prescritto dalla nostra Costituzione.

Ciò eviterà di far regredire il processo ponendo nel nulla attività complesse e costose, innalzando al tempo stesso l'effettività del complessivo sistema delle garanzie. Analogamente, la disciplina delle questioni di competenza deve contemplare rigide preclusioni temporali e l'immediata ricorribilità in Cassazione, piuttosto che la Cassazione torni sul fatto a distanza di anni, in modo da pervenire sul punto ad una rapida e definitiva decisione. Intendo poi (e quando dico «intendo», evidentemente, voglio dire d'intesa con la volontà parlamentare) realizzare una profonda riforma della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge cosiddetta ex Cirielli, così adempiendo ad un preciso impegno di programma. Il cuore dell'intervento deve ancorare il termine finale della prescrizione ad un momento precedente alla formazione del giudicato, evitando la moria dei processi, scoraggiando impugnazioni meramente dilatorie e incentivando il ricorso ai riti alternativi. Va precisato che tale intervento potrà riequilibrare il vigente sistema di inappellabilità della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, pure attualmente sottoposto a vaglio di costituzionalità. Per quanto riguarda i riti alternativi, all'effetto di spinta indotto dalla certezza della conclusione del processo in tempi ragionevoli, vanno affiancate preclusioni temporali al patteggiamento; un patteggiamento ammesso in grado di appello costituisce uno spreco di risorse non giustificato, sicché alla parziale rinuncia dello Stato alla pena deve corrispondere effettivamente un recupero di risorse e di efficienza del sistema. È allo studio inoltre la possibilità dell'allargamento del patteggiamento alle pene, pur non condizionalmente sospese, per le quali l'imputato abbia titolo per l'affidamento in prova al servizio Tale strumento, del quale stiamo verificando il possibile impatto quantitativo, consentirebbe di unificare nella fase preliminare del processo, con evidenti effetti deflattivi, le decisioni relative alla pena da irrogare ed alla sua futura esecuzione. L'intervento, che intendo proporre in uno dei prossimi Consigli dei ministri, comporta altre importanti disposizioni, quali la riforma delle impugnazioni delle misure cautelari e l'archiviazione dei procedimenti per fatti di particolare tenuità. È stato inoltre avviato un qualificato tavolo tecnico per poter varare in tempi brevi un disegno di legge delega in materia antimafia che, coordinando e razionalizzando la normativa esistente, sia diretto a realizzare opportune modifiche del codice penale e di procedura penale e delle connesse leggi speciali, in chiave di accresciuta efficienza della complessiva risposta repressiva al fenomeno mafioso. Siamo alla parte finale (questo è dettato come programma, quindi sono costretto e chiedo scusa ai colleghi; mi tocca per disciplina e per modalità istituzionale), che riguarda la giustizia minorile. In sintonia con i sistemi di giustizia minorile e le politiche giovanili dei Paesi dell'Unione Europea e coerentemente con gli orientamenti del Governo di razionalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, sarà istituito un Centro per la ricerca, la formazione e l'innovazione del Dipartimento per la giustizia minorile. Il centro garantirà la razionalizzazione delle risorse umane ed economiche e si occuperà di sviluppare la ricerca finalizzata ad azioni innovative e interventi di qualità in area tecnico‑operativa, sostenendo e rafforzando le competenze degli operatori che lavorano in ambito minorile e la cooperazione a livello nazionale, europeo e internazionale. Nel contempo, occorre favorire e diffondere la strategia della mediazione penale, fortemente sostenuta dalle istanze europee. Sarà costituita, inoltre, una commissione incaricata di proporre una complessiva riforma ordinamentale, nella prospettiva di riunire in un unico organo tutte le competenze che attengono alla persona, al minore e alla famiglia. Una diversa commissione studierà invece in particolare l'organizzazione del sistema penitenziario minorile. C'è un altro argomento che è apparso all'orizzonte in questo periodo e che vorrei brevemente trattare, quello che riguarda la soglia di età della responsabilità penale. Ritengo cioè che l'abbassamento di tale soglia, pur presente come ipotesi nel dibattito politico (in Francia si discute di questo, Sarkozy ne ha fatto un elemento di impianto all'interno del suo programma, ritenendo che la punibilità prescinda dal reato come tale: la soglia di punibilità non c'entra assolutamente nulla, interessa il reato anche se può essere compiuto da un ragazzo

nei Paesi dove questa soluzione è stata adottata, le evidenze statistiche non ne hanno dimostrato la pertinenza. Altri strumenti, invece, di carattere socio-educativo, mi paiono più congrui rispetto ai bisogni di prevenzione speciale e culturalmente più vicini alla nostra tradizione giuridica e alla migliore prassi dei nostri uffici giudiziari. Sono poi a parlarvi delle misure di organizzazione, razionalizzazione ed assorbimento dell'arretrato. Sono tutti interventi, questi, necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Non si può immaginare o (qualcuno) sorridere su questo immaginifico di cinque anni se non si smaltisce l'arretrato. Di particolare rilievo da questo punto di vista è la realizzazione dell'ufficio per il processo, inteso come struttura amministrativa di supporto all'attività giudiziaria. La piena attuazione dei princìpi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata richiede una nuova metodologia di organizzazione del lavoro del personale dell'amministrazione giudiziaria, orientata alle moderne prospettive di lavoro di gruppo e al raggiungimento di obiettivi di efficienza. Il nuovo modello organizzativo proposto è una specie di contenitore flessibile delle diverse professionalità, idoneo quindi a rispondere alle esigenze di ammodernamento, attraverso lo sviluppo della collaborazione e delle sinergie possibili, cioè risorse umane,

Faccio presente che il mio Ministero è uno dei pochi, anzi l'unico, dove non si è mai realizzata la riqualificazione del personale; l'unico Ministero che non ha svolto un'attività di riqualificazione del personale da anni e anni a questa parte. Si tratta quindi di un cronico elemento di disparità anche rispetto agli altri Ministeri. Ministeri. Questo disegno di legge è sviluppato in un'ottica di dialogo con gli operatori del settore e di concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e si propone come intervento normativo quadro di definizione dei princìpi generali della riorganizzazione. L'ufficio per il processo garantisce il compimento, debitamente monitorato, delle attività correlate all'attività giurisdizionale, consentendo anche l'occasione, senza oneri per l'amministrazione, di svolgimento presso di esso di attività di tirocinio legale. Una sorta di sperimentazione

che in maniera, secondo alcuni azzardata, ma io ritengo abbastanza verosimile (per questo la propongo alla vostra attenzione), mi permetto di suggerire al Parlamento. L'istituzione dell'ufficio per il processo è accompagnata da un specifico percorso di valorizzazione del personale, ridefinizione delle mansioni, ricollocazione nei rispettivi inquadramenti, anche in relazione al forte impulso che viene impresso al processo telematico. A questo proposito devo dire che siamo arrivati a un passaggio cruciale, che ci consentirà al tempo stesso il definitivo passaggio (scusate il bisticcio di parole) dal supporto cartaceo al collegamento in rete, per arrivare appunto in maniera definitiva al processo telematico. L'informatizzazione degli uffici giudiziari può realizzare un salto di qualità mettendo a frutto le sperimentazioni e i progetti che sono stati condotti (non da me, evidentemente, ma continuo sulla stessa scia) dal Ministero negli uffici giudiziari. La nostra intenzione è di far divenire le esperienze virtuose, condotte in molti uffici da punte di eccellenza in realtà di nicchia, a quotidianità per tutti gli uffici. La prima dimostrazione di ciò è stata la partenza lo scorso dicembre del decreto ingiuntivo telematico con valore legale presso il tribunale di Milano. È nostra intenzione ora estendere questa esperienza da laboratorio in altre sedi in Italia. L'obiettivo è di realizzare entro il 2010 decreti ingiuntivi, notifiche ai legali, processo previdenziale e processo esecutivo in via telematica e con valore legale in tutti gli uffici giudiziari. La realtà più complessa e articolata del processo penale non ha per ora consentito una diffusione così ampia del processo telematico, ma sono in corso sperimentazioni, in particolare per la dematerializzazione e facile consultazione degli atti depositati ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, per la realizzazione della banca dati delle misure cautelari, per il sistema informativo dell'esecuzione penale e per il sistema informativo delle misure di prevenzione personali e reali (i beni confiscati, ad esempio, alla criminalità organizzata). La riforma organizzativa è altresì diretta alla semplificazione delle attività di pagamento di contributi, diritti e spese processuali ed alla razionalizzazione della gestione delle somme confluenti nei depositi giudiziari. Tutto ciò nel quadro di uno sforzo più generale che la mia amministrazione sta assicurando per il contenimento e la razionalizzazione delle spese. In particolare, a proposito delle spese, vengo alla *vexata* *quaestio* delle intercettazioni telefoniche. Appare ineludibile una concorde azione del Governo per modificare sostanzialmente le prestazioni obbligatorie dei gestori di telefonia e correggere, anche per il passato, evidenti distorsioni nei meccanismi e nei risultati di spesa. La spesa per le intercettazioni telefoniche e ambientali è infatti elevatissima. Nel quadriennio 2006-2006 il costo globale è stato di circa 1.300.000.000 euro e in tale somma non è compreso il costo delle trascrizioni. Tali costi sono il risultato di una gestione non centralizzata e del tutto irrazionale, assolutamente non governata nello scorso quinquennio dall'amministrazione centrale. I contratti di nolo degli apparati su base circoscrizionale registrano altissime variazioni dei costi da sede a sede (il ventaglio dei costi va da uno a diciotto). Inoltre, dovrà essere rivista la base di costo fissata con i gestori di telefonia obbligati per legge a fornire la prestazione.

Il costo per spese di investimento, cablaggio, misure di sicurezza dei locali, postazioni informatiche, acquisto *software* e manutenzione è stimato in 19.292.500 euro. All'evidenza è possibile un enorme recupero di risorse (da oltre 300 a circa 20 milioni di euro all'anno). Ma ciò che mi sembra cruciale, onorevoli senatori, è che venga pienamente tutelato il pieno controllo dell'autorità giudiziaria sul dato investigativo, garantendo concretamente l'accessibilità ad uno strumento d'indagine insostituibile nelle indagini più complesse e più delicate. L'efficacia delle nuove norme processuali e organizzative si confronterà però con uno spaventoso arretrato, per il quale vanno realizzati interventi straordinari di abbattimento. Per il civile è possibile procedere con meccanismi di stralcio per la rapida evasione di tutte quelle cause rimaste prive di sufficiente trattazione probatoria che abbiano superato o stiano per superare gli *standard* di ragionevole durata determinati dalla giurisprudenza della Corte europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo. Questa misura straordinaria necessita, per raggiungere rapidamente gli obiettivi di azzeramento dell'arretrato, del reclutamento e retribuzione di magistrati onorari, in ragione di ogni sentenza prodotta. Solo così si garantisce, forse, che la retribuzione sia direttamente collegata al risultato, evitando al contempo future rivendicazioni di stabilizzazione. Per i processi penali l'unica misura allo stato possibile è una norma transitoria che consenta l'applicazione del patteggiamento per reati coperti da indulto con una deroga agli attuali sbarramenti temporali. Si impongono inoltre, in coerenza con gli impegni di programma, le modifiche radicali agli interventi, cosiddetti *ad personam*, in primo luogo in materia di falso in bilancio. In definitiva, come come ho più volte ripetuto, il Ministro della giustizia dev'essere messo in condizione di far fronte alle responsabilità che l'articolo 110 della Costituzione gli attribuisce sull'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Nel contempo,

In tale ottica sono pronto, dunque, alla presentazione nei prossimi giorni e già da oggi dei disegni di legge che vi ho illustrato, attento a valutare ogni ulteriore suggerimento che dovesse giungermi. Cari colleghi, a tutti voi chiedo non una ripartenza, come si dice con linguaggio un po' ferroviario, ma di essere partecipi e protagonisti di una «missione» che alcuni affermano essere improbabile e qualcuno denuncia come impossibile. Sono convinto che la giustizia è rispettata se funziona e noi dobbiamo, anzi abbiamo il dovere etico di farla funzionare. Il principio sacro della indipendenza (che è anche il mio, per la verità), poiché è il cardine di qualunque democrazia, sarà apprezzato e difeso da una larga base sociale, non solo per ragioni fideistiche rispetto a quei valori, ma grazie al fatto che il sistema funziona. Questa è la giustizia che attendono i cittadini.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il discorso programmatico svolto dal Ministro è da apprezzare indica un programma positivo da sostenere e da portare avanti. Vi è anche una novità politica significativa: la volontà del Ministro della giustizia di cambiare le leggi sbagliate della passata legislatura, a partire dal falso in bilancio e dalle leggi *ad personam*. Condividendo l'impianto di fondo della sua proposta, mi limiterò nel mio intervento a dare alcuni suggerimenti, come egli stesso ha chiesto. Innanzitutto, insistere per ottenere adeguati stanziamenti per la giustizia. I numeri che lei ci ha fornito, signor Ministro, sono drammatici e confermano l'aggravarsi di una situazione molto seria. Sono necessari investimenti e risorse per due ragioni. La prima è che il diritto alla giustizia è un diritto costituzionale

che il funzionamento efficace del sistema giustizia fa parte della competitività del sistema Italia. In secondo luogo, vi è il problema dei tempi, non del programma nel suo insieme, insieme, che è ampio, ambizioso e richiede perciò il tempo della legislatura. Vi sono, però, alcune urgenze, alcune anticipazioni delle riforme. Per esempio, il sistema della prescrizione. Io credo che del lavoro meritoriamente svolto dalle Commissioni alcune parti vadano stralciate, anticipate in modo da poter affrontare tempestivamente alcune emergenze. Sono allarmato per i tempi della riforma dell'ordinamento giudiziario. Se non ho inteso male...

Se non ho inteso male, ella, signor Ministro, ci ha detto che oggi è stato diramato il testo della riforma dell'ordinamento giudiziario. Ora siamo molto vicini parlamentarmente alla scadenza di luglio, che ci demmo diversi mesi fa, e bisogna che in Parlamento sia depositato al più presto il disegno di legge del Governo per poter affrontare nel merito le questioni ed evitare una drammatizzazione. Tre suggerimenti, signor Ministro, ancora: sugli effetti dell'indulto, sulla decisione che dovrà essere presa sul caso Abu Omar e sulla discussione che c'è stata, che è in corso in questi giorni, su un preannunciato provvedimento concernente la *Shoah*. Comincio dal primo punto. La legge sull'indulto è alle spalle, ci sono state polemiche che non avrebbe senso riprendere; lei se l'è coraggiosamente intestata, anche se è stata votata, come richiesto dalla Costituzione, da una larga maggioranza del Parlamento. Ora il punto è fatto l'indulto, noi dobbiamo evitare che si riproponga la stessa situazione preesistente all'indulto. La misura era giusta in sé - poi sulle modalità ci sono state opinioni diverse - per rendere le carceri più umane. Le carceri si rendono più umane evitando il sovraffollamento e creando condizioni di vita dignitose per i detenuti; ora le carceri stanno tornando ad affollarsi. Il garante dei diritti dei detenuti di Firenze, Corleone, che ho ricevuto in questi giorni insieme ad altri garanti di detenuti, danno cifre concrete. Nel carcere di Sollicciano prima dell'indulto c'erano mille detenuti; si era passati a 576; ora sono già oltre 700. Perché? Perché ci sono delle leggi che condannano a stare in carcere persone che probabilmente non ci devono stare: e sono gli immigrati extracomunitari che hanno la sola colpa di non essersi allontanati dell'Italia; e c'è quel problema che sappiamo dell'equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere sulla tossicodipendenza. Questo è un punto che va affrontato, altrimenti fra pochi mesi riavremo quel numero e quelle persone che non credo siano le più pericolose per la collettività nazionale, se è vero che il carcere dev'essere l'*extrema* *ratio.* Bisogna, signor Ministro, che nel carcere i detenuti siano trattati civilmente. Segnalo due punti. Anzitutto, la difficoltà ad avere assistenza legale; questo sistema della difesa dei non abbienti e del gratuito patrocinio va fatto funzionare, perché sono proprio queste persone di cui si parlava che non sanno nemmeno come fare funzionare il Ministro della giustizia)* e le condizioni - vero, senatore Ladu? - della salute nelle carceri. Bisogna risolvere questo sistema della doppia amministrazione. Il diritto alla salute, di cui parla la Costituzione, vale per chi sta in carcere come per chi sta in libertà, ma così non è, con problemi molto gravi e molto seri. La seconda questione riguarda il caso Abu Omar. Signor Ministro, c'è un'interrogazione che attende una sua risposta, sottoscritta da esponenti della Commissione giustizia di tutti i Gruppi di centro-sinistra. Noi le chiediamo di sciogliere questo nodo, di scioglierlo rapidamente e di scioglierlo in senso positivo. La richiesta della procura di Milano non è quella non è quella di dichiarare guerra agli Stati Uniti d'America e nemmeno quella di negargli basi militari: la richiesta della procura di Milano è che, sulla base delle indagini che si sono svolte e dopo oltre tutto che ieri una risoluzione dell'Europarlamento ha segnalato la gravità delle operazioni di *extraordinary rendition*, il Governo italiano faccia la sua parte. C'è qualche motivo per cui non si debba chiedere l'estradizione? Non stiamo chiedendo di spedire truppe in missione per catturarle: stiamo chiedendo che il Governo italiano chieda al Governo degli Stati Uniti di mettere a disposizione della giustizia italiana persone che sono processate per un reato gravissimo. Ne va del rispetto della legalità internazionale, ne va della sovranità nazionale e, se permettete, anche della dignità italiana.

La *Shoah* è stata la grande tragedia del '900 europeo e il negazionismo è una vergogna. Proprio per questa ragione (ho visto che lei poi

e perché il negazionismo è una vergogna, dico con chiarezza che noi europei non possiamo pensare di salvarci l'anima di europei limitando la libertà di opinione di qualche emulo del nazismo. La possibilità di esprimere opinioni è una garanzia delle libertà, dei diritti di libertà, che non può essere repressa con leggi. La battaglia contro l'antisemitismo, la battaglia contro il negazionismo, la battaglia contro ogni forma di concezione razzista va condotta con grande impegno culturale e ideale, anche con leggi che rispettino però il principio della libertà di opinione e della libertà di ricerca scientifica. Combattere tutte le forme di intolleranza ed è possibile e necessario: tanto più è possibile farlo se si parte dalla difesa delle istituzioni e delle regole della cultura politica e giuridica liberale. Ho sottolineato questi punti, signor Ministro, proprio perché - come ho detto all'inizio - condivido il programma che è stato predisposto. Per quanto mi riguarda, come Presidente della Commissione giustizia mi auguro che i lavori della Commissione possano procedere come è stato in questi mesi do atto a tutti i colleghi che ne fanno parte, della maggioranza come dell'opposizione - in una dialettica a volte serrata, ma in un grande spirito di collaborazione. Io mi propongo, e tutti noi ci proponiamo, di proseguire in questa direzione. In Senato abbiamo approvato due leggi importanti, sulle intercettazioni e sull'ordinamento giudiziario, seguendo questo metodo. Altre leggi importanti abbiamo al nostro esame: penso che il Parlamento possa - nella doverosa dialettica fra maggioranza e opposizione, ma nello spirito di concordia che è tanto più necessario quando si affronta un problema così rilevante e drammatico come quello della giustizia italiana - collaborare in spirito costruttivo,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, poiché interverrò molto probabilmente anche nella fase delle dichiarazioni di voto per ora mi limito ad alcune osservazioni e anche io, imitando il mio Presidente di Commissione, darò qualche suggerimento. Siamo senz'altro d'accordo su questo suo programma, o per meglio dire su questa sua dichiarazione di intenti che delinea quello che poi sarà il programma del Governo, che saremo in grado di apprezzare quando ci verranno presentati i testi

ha messo in risalto il problema di un monitoraggio del settore giustizia con l'ausilio di tecnici e anche di statistici. Le devo ricordare che il precedente Governo ha bandito un concorso per 40 posti di statistico: tale concorso è stato espletato, i concorrenti vincitori si sono visti pubblicare il nome sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma da anni attendono di essere chiamati. Credo che questa sia una buona occasione, non solo per chiamarli tutti, ma anche per far scorrere la graduatoria.

e programmaticamente è un *déjà vu*, una cosa già vista, perché si tratta di sfidare le leggi della matematica.

quando al dibattimento o all'udienza arriva con un mare di fascicoli e non è in grado nemmeno di fissare l'udienza ad un anno. Quindi, bisogna affrontare questo problema con coraggio, ma anche disponendo di risorse.

ma mantenere ferma la validità della non appellabilità della sentenza di assoluzione in primo grado, quando essa sia però una assoluzione dibattimentale limitata all'assoluzione con la vecchia formula piena, cioè quando l'imputato non ha commesso il fatto o il fatto non sussiste. sussiste. Dare il crisma dell'inappellabilità anche all'archiviazione mi sembra qualcosa che va contro, non solo la nostra tradizione giuridica, ma anche la logica. Quindi, manteniamo fermo questo pilastro: l'assoluzione in primo grado con formula piena diventa inappellabile, ovviamente ricorribile in Cassazione perché c'è la Costituzione che lo impone. Un altro suggerimento è quello di pensare bene all'ordinamento giudiziario, agli attori in campo,

Non c'è dubbio che il tema fondamentale di scontro tra magistrati e avvocati è quello della separazione delle carriere e non c'è dubbio che nel nostro programma elettorale tale separazione non è prevista; c'è un impegno per la distinzione. Però, siccome il contrasto rimarrà e noi dobbiamo assolutamente far sì che esso si affievolisca il più possibile, anche la distinzione delle funzioni va applicata seriamente:

perché all'interno del distretto c'è questo gioco di poltrone: il capo dei gip diventa presidente del tribunale, il presidente del tribunale va a fare il procuratore della Repubblica, il procuratore della Repubblica va a fare il procuratore generale, nel frattempo il procuratore generale va a fare il presidente della corte d'appello, con un vorticoso giro di poltrone che rende il potere giudiziario in quel distretto

non irritare ulteriormente gli avvocati, dobbiamo far sì che questa distinzione delle funzioni sia seria e che lo sia anche in relazione ai distretti.

Peraltro, lo dicevo anche quando abbiamo realizzato quella grande riforma della prima parte dell'ordinamento giudiziario, non c'è dubbio che dobbiamo avere una riforma condivisa perché solo così l'ordinamento giudiziario e le leggi ulteriori che verranno saranno più apprezzate dai cittadini, più condivise. Perché un ordinamento giudiziario ha la sua forza proprio nella condivisione: l'ordinamento giudiziario inglese o francese è un ordinamento che i cittadini stessi condividono, anche perché poi lì (specialmente in Inghilterra) le cause penali durano pochissimo. Ma, ripeto, il sistema in sé è un sistema che

trovare un'intesa con l'opposizione. Come lei, signor Ministro, ha giustamente e saggiamente operato nella riforma dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e del disciplinare, così dobbiamo, con quello stesso intento riformatore, andare avanti perché in quella fase abbiamo trovato un'opposizione che ha recepito in pieno

Signor Presidente del Senato, signor Ministro, signori senatori, il testo della relazione del Guardasigilli sull'amministrazione della giustizia si è proposto di delineare i tratti principali dei progetti di riforma che il Ministro stesso ha intenzione di presentare al Consiglio dei ministri. Questa relazione fotografa molto bene lo stato della giustizia in Italia: il tratto più evidente e più grave è quello della insoddisfazione dei cittadini verso l'insieme del sistema giustizia. Quello che la relazione del Ministro non fa, e non può forse fare in questa fase, è il tentativo di individuare la causa, o meglio le cause, di tale profonda insoddisfazione. Quando mi capita, un po' in tutta Italia, di partecipare ad incontri con i cittadini su questa tematica rilevo che due sono le questioni fondamentali che vengono poste: quella dei tempi dei processi e quella della certezza della pena. Un cittadino che si trova per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo ad avere a che fare con i tribunali sa bene quando inizia, ma non sa quando finirà; i processi iniziano sempre, ma rischiano di non finire mai. I dati forniti dal Ministero, peraltro noti almeno in parte, vengono a confermare l'osservazione di questo stato pressoché fallimentare, quasi da bancarotta. Durante i lavori della Commissione giustizia in ordine alla discussione della legge finanziaria, praticamente tutti i senatori intervenuti hanno dovuto rilevare il *trend* sostanzialmente negativo nel bilancio pubblico delle spese relative al comparto giustizia concernenti il personale fisso e precario, le strutture edilizie, i mezzi necessari per far funzionare la macchina della giustizia, l'informatizzazione degli uffici giudiziari. La Commissione in quella fase, pur esprimendo una fortissima preoccupazione, apriva una linea di credito a favore del Governo in un'ottica complessiva di risanamento delle finanze e del bilancio pubblici, ma esprimendo la speranza di una maggiore attenzione per i problemi della giustizia, della quale, come ha ben detto il ministro Mastella, va affermata la centralità quale vero pilastro dell'ordinamento democratico a tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini. Ora, in questo momento, dopo aver fotografato la gravità della situazione, il Ministro propone delle linee di intervento e prospetta dei disegni di legge. Se ritengo, come ritengo, di condividere pressoché totalmente fotografia, proposte e prospettazioni del Ministro, non posso non rilevare che, al momento, è chiesta l'apertura di un'altra linea di credito. Il fatto è che noi della maggioranza non possiamo presentarci al Paese come coloro che hanno fatto l'indulto, provvedimento che pure ho condiviso e votato e non rinnego assolutamente. All'interno del nostro programma elettorale, in materia di giustizia, si trovano proposte concrete e specifiche, che sono poi quelle riprese nella relazione odierna del Ministro. Così come rappresentate, non possono che essere condivise, purché siano realmente sostenute e portate avanti in ogni sede competente. È giusta la preoccupazione del Ministro di pensare ai costi della giustizia, è ancora più importante pensare a rendere più efficaci gli interventi e più efficiente la macchina. Il piano straordinario di interventi proposto dal Ministro individua esattamente i settori per così dire dolenti: l'ordinamento giudiziario, il processo penale e civile, le misure di riorganizzazione e razionalizzazione, la correzione delle norme cosiddette *ad* *personam*. Per evidenti ragioni di tempo mi limito a toccare qualche punto. Sull'ordinamento giudiziario, aspettiamo il testo del Governo, rammentando vivamente che il disegno di legge va approvato da entrambi i rami del Parlamento entro il 31 luglio del 2007. Gli interventi proposti in ordine a riforme del processo sia civile che penale, se realmente portati avanti e fatti giungere in porto, si presentano, a mio parere, come sicuramente idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati: deflazione e tempi ragionevoli per la durata dei processi. Credo, peraltro, che sia giunto il momento di pensare anche ad una diminuzione, o comunque ad una reimpostazione, dei vari gradi di giudizio che certamente contribuiscono ad una proliferazione processuale e ad una dilatazione dei tempi, inesistenti in qualsiasi altro Stato estero. Al di là delle specifiche proposte illustrate dal Ministro, ritengo veramente fondamentale che arrivino finalmente a conclusione i lavori delle commissioni ministeriali in materia di codice penale e di codice di rito penale,

al riguardo, alle perplessità già indicate in premessa per quanto attiene alla necessità e all'inderogabilità di un serio impegno finanziario proprio per consentire un rapido passaggio dal supporto processuale cartaceo al collegamento in rete con la finalità di giungere ad un processo di natura telematica. In materia di intercettazioni telefoniche, mi rifarei sinteticamente alle conclusioni dell'inchiesta svolta di recente dalla Commissione giustizia per quanto concerne sia gli aspetti di necessità per le indagini di questo strumento investigativo, sia il delicato tema della tutela e del rispetto della persona e della *privacy*, sia il problema dei costi. Problema dei costi da affrontare sotto una triplice angolatura: formazione dei capi degli uffici giudiziari in ottica manageriale; controllo dei costi delle apparecchiature, secondo quanto prospettato anche dal Ministro nella revisione dei rapporti finanziari con le società di gestione di telefonia, mirando o al modello germanico o ad una forfetizzazione dei costi. Voglio riservare la parte conclusiva del mio intervento ad uno dei punti toccati anche dalla relazione del Ministro, la questione dell'abrogazione o, comunque, della profonda modifica delle leggi cosiddette *ad personam*, eredità infausta del precedente Governo. Non ci si può limitare ad un semplice accenno, anche perché il tema della legalità è uno dei più fortemente vissuti e sentiti dalla nostra gente. Nel programma elettorale avevamo inserito chiaramente la volontà di abrogare tali leggi (la ex Cirielli, la Cirami e quella sul falso in bilancio), ora non possiamo far finta di nulla: come senatori dell'Ulivo, abbiamo presentato da tempo disegni di legge in materia, di cui si occuperà la Commissione giustizia del Senato; sarebbe, però, molto utile e confortante un intervento chiaro, dettagliato e preciso, a questo proposito, anche da parte dei Governi. concludere: il contenuto della relazione del Ministro non può che essere pienamente condiviso; l'auspicio - la speranza - è che le proposte del Governo si concretizzino al più presto.

mi ero formato l'idea che i giornalisti avessero mal compreso il suo discorso e che i loro resoconti fossero errati. Dall'esito di un difficile ascolto della sua relazione, mi rendo conto, invece, che la mia era un'idea sbagliata, o meglio: sicuramente i giornalisti hanno, per così dire, mal riportato il senso del suo intervento, ma per difetto; a cominciare, ad esempio, dal fatto, signor Ministro, che lei, sia pur con maggior garbo e simpatia, ci è venuto a ripetere quanto nella scorsa legislatura in Commissione ci veniva detto da Edmondo Bruti Liberati, all'epoca presidente dell'Associazione nazionale magistrati. In altri termini, signor Ministro, ho la forte impressione che lei, forse tradendo - come dire? - la sua funzione, abbia compiuto una scelta di campo: si è appiattito sulle posizioni dell'Associazione nazionale magistrati. Ha affermato - se è vero quanto ho letto sul giornale - che questa è una scommessa: mi permetto di ricordarle che le scommesse si fanno, se si vuole, alle corse dei cavalli, ma che, in sede legislativa, dovrebbero essere evitate, in quanto la legge dovrebbe essere il frutto di un serio approfondimento e di una seria programmazione.

lei non ha dedicato una sola parola al sistema penitenziario, dicevo, e questo è davvero molto grave, se si pensa che solo qualche mese fa il Parlamento ha varato una legge sull'indulto che si fondava proprio sulla difficoltà del sistema penitenziario. Allora, volevamo capire fin da subito quali fossero le sue idee sul punto, per non doverci trovare, di qui a qualche anno, di nuovo costretti, per l'inefficienza del sistema penitenziario, a varare una nuova legge sull'indulto. Nel corso del suo intervento lei ha toccato vari punti, ed evidentemente per ragioni di tempo non potrò che dedicare la mia attenzione solo a taluni di essi. Il primo: lei ha definito la procedura dell'ordinamento giudiziario Castelli per la valutazione dei magistrati una procedura bizantina, dimenticando, però, che i criteri di valutazione previsti in quell'ordinamento giudiziario erano tutti centrati sull'attività e sulla professionalità dei magistrati e ci dice, sostanzialmente, che è nella sua idea immaginare una valutazione ogni quattro anni dell'attività e della professionalità del magistrato. Ma lo sa o non lo sa, signor Ministro, che il magistrato viene valutato normalmente dopo un anno, dopo cinque anni, dopo tredici anni, dopo vent'anni e dopo ventisette anni e che non vi è un solo rapporto negativo nei confronti dei magistrati? I magistrati sono l'unica categoria che ha la caratteristica di essere rappresentata da uomini eccezionali; questo è quello che dicono i loro rapporti. E poi, signor Ministro, è troppo facile dire «ogni quattro anni valutiamo il magistrato»: chi lo valuta, il magistrato? Il Consiglio giudiziario, e cioè nuovamente una consorteria associativa, sì che eventualmente un magistrato che voglia cantare fuori dal coro può trovarsi esposto ad una valutazione di tipo negativo? Ancora: lei parla di una carriera unica, ma era carriera unica anche nell'ordinamento giudiziario Castelli, e ci dice, ma questo già lo rilevava il senatore Di Lello Finuoli, che la sua idea è quella di immaginare che un magistrato che voglia passare dalla funzione giudicante alla funzione requirente o viceversa debba frequentare un corso di formazione, debba essere sottoposto ad un giudizio di idoneità specifica; ma lo sa o non lo sa, signor Ministro, che questo giudizio di idoneità specifica è già previsto nell'attuale normativa consiliare, sia per il passaggio delle funzioni e sia anche - lo dico così, tanto per dirlo - per l'assunzione delle funzioni di legittimità? E lo sa o non lo sa, signor Ministro, che non vi è stata una sola pronuncia negativa sulla specifica idoneità al passaggio delle funzioni o sulla idoneità ad assumere le funzioni di legittimità? In altri termini, lo sa o non lo sa, signor Ministro, che quello che immagina lei per la valutazione della professionalità dei magistrati non garantirà che i migliori «andranno avanti», ma garantirà semplicemente la persistenza di un sistema anomalo e per certi versi perverso, dove ad andare avanti saranno solo gli amici delle correnti o quelli che godono di particolari frequentazioni salottiere? Ancora, signor Ministro: lei parla di una motivazione non sovrabbondante come uno dei criteri per velocizzare il processo e sostituire quella motivazione con una motivazione succinta. Benissimo, ma allora mi vuole spiegare lei come verrà valutata la professionalità dei magistrati se l'apporto di conoscenza giuridica proprio di una motivazione viene meno per essere la motivazione stessa diventata succinta? E ancora, signor Ministro (con molta rapidità, perché il tempo è davvero poco): la durata dei processi sarà di cinque anni;

Come fa, signor Ministro, ad immaginare che un processo possa durare cinque anni quando, ad esempio, per determinati reati - e non parlo di quelli di terrorismo e di criminalità organizzata, per i quali lei ha immaginato un percorso diverso è previsto, che in fase istruttoria l'indagine possa durare un anno e otto mesi. Come fa, signor Ministro, ad immaginare, non esistendo soltanto il reato di associazione mafiosa e di traffico di stupefacenti ma anche quello di associazione a delinquere, che un cosiddetto maxiprocesso possa essere smaltito in fase dibattimentale nei ristretti termini che lei immagina?

in ordine alla depenalizzazione e ai tempi della riforma del codice penale, cioè in ordine alle riforme degli strumenti codice sostanziale e codice procedurale, che sono necessari - questi sì per la riduzione dei termini dei processi, ai quali sicuramente - lo dico con molta franchezza - non gioverà l'altra affermazione propagandistica in base alla quale i magistrati invece di avere quarantacinque giorni di ferie,

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, da troppo tempo nel nostro Paese si parla della giustizia come di un problema. Sicuramente i cinque anni di Governo di centro-destra hanno lasciato un'eredità pesante in questo senso, ma non credo che il centro-sinistra possa liquidare la discussione semplicemente attribuendo colpe a chi ha governato prima. Sarebbe inutile e riduttivo. C'è una incapacità sistemica a risolvere i problemi della giustizia. C'è una difficoltà a liberarsi da vecchi stereotipi per legiferare su un sistema in crisi. C'è una mancanza di equilibrio, una crisi di equilibrio che è diventata crisi politica. Credo che lo sforzo che si deve fare all'inizio di una nuova legislatura sia quello di affrontare il problema come un problema di sistema, del sistema-giustizia all'interno di un problema di organizzazione politica dello Stato, uno Stato che ancora non ha trovato un suo assetto definitivo e che ancora viene definito con il termine «transizione». Abbiamo un sistema politico bipolare, un bipolarismo pieno di contraddizioni, con oltre venti partiti, alcuni dei quali fanno ancora fatica a superare l'approccio ideologico tipico di un sistema proporzionale. Questa giustizia è figlia di quelle contraddizioni. Nell'era del bipolarismo l'approccio dovrà essere quello della risoluzione dei problemi a partire dai bisogni del cittadino, che poi non è altro che la stessa persona che l'economia chiama consumatore e che la politica chiama elettorato. Ancora; dovremo affrontare il problema senza avere atteggiamenti punitivi nei confronti della magistratura, ma anche senza riconoscere ad essa, pregiudizialmente, una delega in bianco. Abbiamo già sperimentato nelle scorse legislature come questo approccio non abbia aiutato a risolvere i problemi della giustizia, anzi sia servito solo ad aggravare la competizione tra i vari operatori del settore a discapito dei cittadini, che sono spesso rimasti con una sensazione di impotenza o, nel migliore dei casi, come dice il Ministro, di rabbia nei confronti dello Stato. Ogni approccio correttivo dovrà partire da una visione di sistema. Quindi non interventi occasionali, ma interventi che affrontino i problemi alla radice, interventi capaci di modificare il quadro, innovando contenuti e metodi. contenuti e metodi. È questo il compito della politica. Oggi, credo, ognuno di noi sa quello che non vuole, quello che bisogna assolutamente cambiare. Dobbiamo andare oltre; dobbiamo essere capaci, in questa legislatura, di ripensare alla giustizia nel suo complesso, a partire dalla risoluzione di problemi ormai evidenti, sapendo però che non basta a questo settore modificare qualcosina; anzi, modificare qualcosa senza intervenire sul tutto, nel mondo del diritto, crea maggiori squilibri di quanti se ne vogliano evitare. Ormai è chiaro, soprattutto alla luce della dialettica molto aspra che c'è stata in questi anni, che non c'è una verità da tutelare e da difendere. E' l'intero sistema in crisi: una magistratura che si sente aggredita, un'avvocatura poco disponibile a ripensarsi fuori da vecchi schemi, un mondo legato all'amministrazione che fa fatica ad adattarsi a tecniche e a modalità operative più efficienti. Riassumendo, potremmo dire: ognuno gioca in difesa; non possono però giocare in difesa gli utenti della giustizia, che, o perché parti offese o perché imputati, si trovano obbligati a far uso di questo strumento per la risoluzione dei loro problemi. In questi giorni stiamo discutendo provvedimenti importanti, Ministro: i diritti da riconoscere alle coppie di fatto, una nuova identità anagrafica attraverso la possibilità anche per la donna di trasmettere il proprio cognome ai figli, il problema del disagio abitativo e degli sfratti, una nuova normativa sulle violenze domestiche; c'è molta carne al fuoco, ma credo che una legislazione su questi temi, anche se buona, magari sarà utile a risolvere alcune lacune legislative, ma non basterà a risolvere i problemi del mondo della giustizia, perché questi sono problemi strutturali. C'è bisogno di ripensare alla quantità e alla qualità degli avvocati; alla quantità, qualità ed efficienza dei giudici. Abbiamo bisogno di una classe forense più competitiva che non lavori su rendite di posizione. Abbiamo bisogno che il Consiglio superiore della magistratura funzioni in modo assolutamente diverso. Dobbiamo riformare il codice penale e rimettere mano alla procedura: da troppi anni si nominano commissioni per progetti che poi non vengono mai portati all'approvazione del Parlamento. Abbiamo bisogno di poter dare voce alle parti offese dai reati. Abbiamo bisogno di maggiori garanzie per l'imputato, per la sua *privacy.* Abbiamo bisogno di una nuova normativa - anche questa più a tutela del cittadino - per i reati di diffamazione a mezzo stampa o di calunnia. C'è bisogno, soprattutto, di un intervento decisivo che incida sui tempi ancora troppo lunghi dei processi, che snellisca i passaggi della procedura penale senza cedere sulle garanzie, che cancelli i tempi morti dei processi civili senza ostacolare un serio accertamento della verità. C'è bisogno di ripensare la riforma dell'ordinamento giudiziario, con un'impronta che non sia ingiustificatamente punitiva nei confronti dei magistrati, ma che contenga regole capaci di portare ad un sistema più giusto. Per questo non c'è bisogno, ad esempio, di una netta separazione delle carriere se è vera e senza eccezioni la separazione delle funzioni; non è necessario impedire o limitare a dismisura il passaggio di funzioni se è ferma la norma che impone, ad esempio, di esercitare le nuove funzioni in un diverso circondario. Va ripensata con attenzione la gerarchizzazione degli uffici della procura. È necessario rivedere i criteri per la progressione dei giudici in carriera, che deve essere legata a princìpi di valore e di efficienza. Più in generale, occorre un serio sistema di verifiche e di controlli sulla qualità e sulla quantità, attribuendo magari in questo senso un reale potere ai consigli giudiziari. Sono d'accordo, signor Ministro, con l'impostazione della sua relazione. Mi auguro che ci sia la possibilità di preparare tali modifiche sostanziali del sistema giustizia, favorendo un ampio dibattito dentro e fuori il Parlamento.

ho ascoltato con molta attenzione ed estremo interesse la sua relazione, nella mia duplice veste di parlamentare e di avvocato. Devo ricordarle, poiché non pretendo che ne conservi memoria, che in Commissione, allorquando lei illustrò le sue linee programmatiche, io dichiarai immediatamente la mia disponibilità rispetto a un percorso di confronto responsabile sui temi della giustizia. Non le nascondo oggi la mia profonda delusione rispetto al cambiamento di rotta evidenziato nella sua relazione. Non ho infatti ascoltato nel corso della sua relazione alcuna valutazione circa i veri problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia e non ho ascoltato alcunché in ordine alla volontà del Governo di procedere a scelte definitive e coraggiose che possano ricondurre alla normalità quel rapporto tra cittadino e giustizia totalmente deteriorato, al punto che, come lei stesso afferma, la stragrande maggioranza dei consociati non ripone più alcuna fiducia nella risposta giudiziaria in questo Paese. Le scelte coraggiose rispetto alla modernizzazione del sistema e al suo recupero di credibilità non consistono certamente nel ricorso da lei annunciato al compromesso della distinzione delle funzioni tra magistratura requirente e giudicante, soltanto demagogicamente tesa alla difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, ma in realtà orientata alla conservazione di antichi e ormai anacronistici privilegi.

ha sostenuto giustamente che non vi può essere terzietà effettiva e sostanziale del giudice (dunque piena applicazione dei princìpi dell'articolo 111 della Costituzione) se non si realizza la separazione delle carriere e, ancora, che non vi può essere, sempre in ossequio al medesimo precetto costituzionale, parità tra accusa e difesa nel processo penale senza un'effettiva separazione delle carriere giudicanti e requirenti. Non so proprio come farete voi della maggioranza a conciliare queste diverse posizioni distinte e distanti, che finiranno poi per provocare dei chiarimenti che potrebbero condurre all'esplosione di questa maggioranza. c'è un'ipocrisia di fondo

signor Ministro, c'è un'ipocrisia di fondo nell'approccio che il potere politico continua ad avere quando affronta l'emergenza giustizia nel nostro Paese. Mi auguravo che lei la superasse ma mi accorgo che evidentemente Questa ipocrisia di fondo porta a bloccare l'analisi dei problemi agli aspetti strutturali e a quelli normativi, facendo finta di non sapere che esiste anche e soprattutto un problema umano. Non è un problema di norme, ma è un problema soprattutto di uomini. Esiste in questo Paese soprattutto il problema del chi e del come amministra la giustizia. Esiste il problema degli abusi e delle forzature che impunemente della legge compie chi è chiamato ad applicarla e a rispettarla. E non si risponda a questo mio tentativo di uscire dall'ipocrisia istituzionale che caratterizza ormai il dibattito sulla giustizia accusandomi magari di muovere un attacco preconcetto alla magistratura; non è così. Mi onoro di avere ottimi rapporti di reciproca stima e anche amicali con molti magistrati e da loro raccolgo sempre più spesso l'amarezza per una delegittimazione che spesso muove dall'interno dell'ordine giudiziario e si concretizza in atteggiamenti superficiali ciarlieri, non ortodossi, sganciati da ogni deontologia professionale e persino da ogni legalità. Proprio dalla riflessione offertami da alcuni di questi magistrati muovo per evidenziare come in questo Paese, davanti agli abusi e alle violazioni commessi da alcuni magistrati, si è reagito, non già rimuovendo tali magistrati a seguito di tempestive attività ispettive, ma cambiando la norma, adattandola alle esigenze di colui che l'ha violata e facendo scattare il meccanismo protezionistico dell'appartenenza correntizia, anche in sede disciplinare. Di cambiamento in cambiamento, alla fine abbiamo ottenuto norme, soprattutto in campo penale, in quello della legislazione antimafia in particolare, che ormai scontentano tutti, non garantendo né la libertà, né l'onorabilità del cittadino, né il giusto processo e ancor meno la repressione della criminalità mafiosa. Infatti, ministro Mastella, il cittadino massacrato dalla gogna mediatica, cui viene sottoposto in relazione all'avvio di un'indagine penale, con la conseguente distruzione della sua immagine e della sua dignità, seguita, nella maggioranza dei casi, da pronuncia di proscioglimento, si chiede perché l'autore dell'errore di valutazione, laddove si accertano responsabilità ineludibili, non sia chiamato a risponderne. Di tutto questo e di problemi quotidiani non trovo traccia né accenno nella sua relazione. Prima di concludere - me lo consenta, signor Ministro, con l'amicizia che le ho sempre tributato e la grande stima che le porto vorrei affidarle le ragioni della mia delusione per il suo intervento, anche in qualità di senatore della Calabria. La mia terra a giorni alterni - come tutti sanno è figlia prediletta del suo Governo o madre di tutte le emergenze, ma solo nei dibattiti sulla stampa, perché dagli atti concreti la Calabria sparisce, com'è sparita - lo rilevava oggi un acuto giornalista di un noto quotidiano calabrese - dalla sua relazione. Le chiedo dov'è finito il cosiddetto decreto Locri che ha annunciato per potenziare gli organici di quel distretto giudiziario che più di altri ha bisogno di misure urgenti e straordinarie. Disse di averlo concordato finanche con il Capo dello Stato - di ciò non dubito - ma non ne abbiamo più traccia; anzi, abbiamo prova di un arretramento, visto che proprio a Locri, da oltre un anno, resta scoperto il posto di presidente della corte di assise che dovrebbe addirittura celebrare il processo per l'omicidio del vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Fortugno. Come spiegare ancora che la figlia prediletta dal suo Governo, anziché ricevere aiuto e sostegno in termini concreti, al fine di riaffermare la presenza dello Stato e dei suoi presìdi, venga spogliata della Scuola superiore della magistratura, già assegnatale legittimamente dal Governo Berlusconi? che tale sua scelta sia stata accompagnata da una spiegazione convincente e rispettosa delle legittime aspettative, della dignità e dell'intelligenza dei calabresi. Non si tratta di polemiche pretestuose - me lo consenta di considerazioni che costituiscono, in sintesi, la presa d'atto dell'impossibilità di condivisione di un percorso fatto di riforme, rispetto alle quali mi pare difettino totalmente i presupposti che, per all'avvio della legislatura, ella aveva manifestato di voler porre a fondamento della sua azione di Governo. Signor Presidente, debbo dire che questa è un'ottima occasione. Onorevole Ministro, devo innanzitutto dirle che ho molto apprezzato il passaggio della sua relazione con cui praticamente chiede ai senatori di manifestare le proprie convinzioni per migliorare il suo programma di risanamento della nostra giustizia, così come il riferimento che lei ha fatto alla «giustizia ingiusta». Lei ricorderà che ho intitolato proprio così un mio saggio, perché è vero che una giustizia che arriva troppo tardi è sempre ingiusta: è ingiusta per l'innocente, ma anche per il condannato, per il condannato, molto spesso persona diversa da colui che commise il reato per cui è stato condannato e che prova risentimento verso lo Stato.

così come ho apprezzato il suo tentativo di dare ai nostri giudici un ordinamento giudiziario soddisfacente. I punti che lei ha indicato sono da me perfettamente condivisi. Checché ne dicano gli altri, effettivamente per la prima volta viene affrontato il problema di dichiarare decaduti dalla magistratura i magistrati che non sono degni di esercitare questa professione dopo un doppio giudizio negativo.

di una precisazione successiva. Sarà compito del Parlamento, del Senato - in particolare - indicare chi dovrà giudicare i giudici.

Non vi hanno posto rimedio neanche le leggi della precedente legislatura, molte delle quali lei stesso, signor Ministro, ha proposto di abrogare e di modificare. Non credo, però, che i rimedi da lei suggeriti siano sufficienti a ridurre significativamente i tempi di definizione dei processi. I tempi non si riducono, signor Ministro, né fissando delle sanzioni per i giudici che non rispettano i tempi prestabiliti - i famosi cinque anni anni - né incidendo sui tempi di prescrizione: non facciamo come ha fatto la destra che ha ritenuto di ridurre i tempi dei processi riducendo i tempi di prescrizione. Per ridurre i tempi di definizione dei processi bisogna capire dove ha sbagliato il legislatore del 1988 nel nostro codice. A mio avviso, il legislatore del 1988 non ha avuto il coraggio, pur essendosi ispirato ai princìpi del processo accusatorio, di andare fino in fondo.

di abbandonare quegli istituti che erano stati creati esclusivamente e che calzavano benissimo per il processo inquisitorio del codice Rocco del 1930 ma non erano più significativi e non garantivano più i cittadini per un processo di tipo accusatorio. Signor Ministro, il codice del 1988 ha lasciato praticamente immutato il sistema delle impugnazioni. Il sistema dell'appello e del ricorso per Cassazione è lo stesso del codice Rocco. In più, come lei ha ben notato, vi è il patteggiamento in appello, una cosa

nel processo inquisitorio, il ricorso in appello e poi per Cassazione con la possibilità - ammettiamolo - anche da parte della Cassazione di entrare nel merito (possibilità poi esasperata dalla legge Pecorella) avevano ragion d'essere nel processo in cui la difesa non partecipava alla raccolta della prova, che avveniva, come lei ricorderà certamente, durante l'istruttoria. Ma che senso ha oggi mantenere questi mezzi di impugnazione, quando noi abbiamo introdotto nella nostra Costituzione, modificando l'articolo 111, i princìpi fondamentali del processo accusatorio? Abbiamo stabilito in quell'articolo che la prova deve essere raccolta in contraddittorio tra le parti, su un piano di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. terzo ed imparziale. In riferimento a quello che ha detto prima il senatore Pittelli, un giudice terzo e imparziale - l'ha definito già la Comunità Europea - è terzo e imparziale per tutti gli altri Stati, è il giudice che non ha in alcun modo esaminato la situazione che è chiamato a giudicare, non è un giudice separato. Che cosa bisogna fare allora per accelerare il processo? Si è parlato sempre di certezza del diritto. La prima cosa da fare è quella di restituire alla Cassazione il mero giudizio di legittimità:

Vogliamo pretendere che effettivamente il giudice di appello, che non ha visto raccogliere la prova e che non ha sentito i testimoni, possa giudicare meglio del giudice che invece la nostra Costituzione vuole che assista alla raccolta della prova? Questa è una contraddizione enorme, questo va contro la nostra Costituzione e per cui, siccome vedo che il mio tempo è già finito, una raccomandazione che io le rivolgo è di pensare seriamente ad una riforma del nostro sistema di impugnazione, perché essa ridurrebbe effettivamente e concretamente i tempi di definizione dei processi.

di mancato pignoramento di un ufficiale giudiziario di Verona, forse già famoso, ma che comunque mi introduce nella riflessione: «Si restituisce l'atto inevaso significando non è stato possibile procedere esecutivamente per grave carenza di personale. Su 16 ufficiali giudiziari addetti alle esecuzioni previsti dalla pianta organica ne prestano servizio di fatto solo cinque, di cui uno in *part time* al 50 A tali ufficiali giudiziari superstiti, inoltre, è stato affidato il compito di seguire le esecuzioni anche nel territorio circoscrizionale del tribunale di Legnago ove non è in servizio nessuno dei quattro ufficiali giudiziari previsti. Abbiamo informato della gravità della questione tutti gli uffici gerarchicamente superiori e abbiamo chiesto al signor Ministro e al signor Presidente della Corte una rapida soluzione del problema, ma sinora senza alcun riscontro. Siamo consapevoli che lo stato di dissesto penalizza soprattutto i signori avvocati e in genere gli utenti della giustizia. Siamo altrettanto consapevoli però che il nostro impegno in questo momento è altissimo; confidiamo perciò nella sua comprensione e se è possibile in un suo intervento presso tutti coloro che potrebbero risolvere il problema. (...) Veramente rammaricati per la situazione creatasi e per il disagio che la stessa sta causandole, restiamo a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti». Si tratta di un verbale di pignoramento che ha qualche anno e quindi non si rivolge all'attuale Ministro di competenza.

in Italia e ha riferimento non tanto all'attività giurisdizionale prestata direttamente dai magistrati, ma agli ausiliari della giustizia. Ciò per dire che il problema della giustizia in Italia è veramente drammatico perché

impegnati quelli che riteniamo i diretti protagonisti del dare giustizia, ossia i magistrati e gli avvocati. Potrei però fare un altro esempio persino più concreto, che ancora non ho sentito citare in quest'Aula. I sindaci della mia provincia - non conosco la situazione delle altre province - in questo momento sono molto a disagio, perché quando una ditta vince un appalto è necessario che l'ufficio tecnico del Comune acquisisca una serie di documenti prima di certificare l'avvenuta assegnazione e dare il via quindi ai lavori: tra questi documenti bisogna acquisire anche il certificato

dunque perché il 25 ottobre scorso si è tenuta la giornata europea della giustizia civile e l'Italia ancora una volta si è presentata «a testa bassa». All' inizio di ottobre il Consiglio d'Europa ha denunciato che le deficienze strutturali del sistema giudiziario italiano tali da minacciare lo Stato di diritto. Perché esse sono tali da minacciare lo Stato di diritto? L'ho già detto in altra occasione in questa sede: paradossalmente ci sono funzioni che lo Stato potrebbe,

il problema della giustizia civile dovrebbe essere considerato, non solo da adesso ma ormai da tanti anni, un' emergenza nazionale. Il Governo dovrebbe mobilitare tutte le risorse umane e finanziarie possibili per affrontare il problema seriamente, organicamente e sul piano della concretezza. L'opposizione, di fronte a riforme di così grande importanza, miranti al ripristino della legalità perduta, dovrebbe dare una mano per costruire finalmente un processo che consenta ai cittadini bisognosi di giustizia di rivolgersi allo Stato per ottenerla,

Sarebbe indispensabile un maggior coordinamento e soprattutto uno sforzo di tutti, non solo del Governo e del Parlamento, ma anche della magistratura, dell'avvocatura e di tutti coloro che gravitano nel «sistema giustizia».

forte, idoneo a restituire ai cittadini quella fiducia nella giustizia che oggi è fortemente contestata, potremo ripristinare il principio di legalità indispensabile per la civile convivenza. Non c'è comunque solo un problema di civile convivenza, di fondamento stesso della convivenza all'interno dello Stato: c'è anche il problema di garantire competitività al nostro sistema economico. Justice* (CEPEJ) pubblicato all'inizio di ottobre mostra che le risorse pubbliche impegnate nel settore giustizia in Italia non sono scarse, ma in linea con la media di altri Paesi dell'Europa a 15 che, però, hanno tempi dei processi di molto inferiori; non è in una carenza di spesa la radice dell'inefficienza della nostra macchina giudiziaria. Questa affermazione apparirebbe in contrasto con l'esperienza comune: si porta spesso all'attenzione pubblica il fatto che i tribunali non hanno risorse, al punto da rendere critico anche lo svolgimento dell'attività quotidiana;

La componente incomprimibile della spesa per l'Italia è molto alta: il 77 per cento del *budget* dei tribunali è assorbito dalle retribuzioni dei magistrati e del resto del personale, mentre per esempio in Austria questo rapporto è del 55 per cento, per la Francia del 54 per cento, per Germania e Svezia del 60 Differenze importanti si riscontrano anche nel livello degli stipendi dei magistrati: mentre all'inizio della carriera la retribuzione dei nostri giudici è del tutto in linea con quella degli altri Paesi, non è così per i livelli più alti. Infatti, fatta eccezione per la Svezia, rappresentiamo il caso in cui la progressione di stipendio con l'avanzare della carriera dal livello iniziale a quelli del grado più alto è maggiore: 3,2 volte contro il 2,4 dell'Austria, il 2,2 della Germania e l'1,7 dei Paesi Bassi. Inoltre, il fatto che tale progressione in Italia avvenga per anzianità e non per incarichi svolti fa sì che la platea di soggetti che ne fruisce sia ampia. Le soluzioni per incrementare l'efficienza, dal lato dell'offerta, vanno dunque forse cercate più in una razionalizzazione della spesa e dell'organizzazione generale del settore, che in un aumento della quantità di risorse da impegnare. Alcune disposizioni contenute nella finanziaria

non seleziona in alcun modo l'efficienza del servizio. Ritengo che si possa fare molto da questo punto di vista nella riorganizzazione generale dei tribunali. Il Ministero della giustizia sembra intenda operare tagli e accorpamenti in modo che tutte le strutture giudiziarie contino su un organico minimo di 14 magistrati. Credo che si tratti di un intervento necessario; qualcuno afferma che è contenuto nella misura, però ha già sollevato proteste vivaci. Da alcune analisi econometriche della Commissione tecnica della spesa pubblica e dell'ISAE sembrerebbe però che per il sistema italiano sarebbe ottimale un minimo di 20 magistrati per tribunale, mentre il 72 per cento dei tribunali è attualmente sottodimensionato e, in passato, le *performance* della giustizia sono migliorate in occasione di riforme che hanno aumentato la dimensione media dei tribunali.

della risposta di giustizia e quindi alla formazione e valutazione dell'attività dei magistrati, che, ovviamente, va calibrata in funzione di un'efficienza

che, senza essere osteggiate dall'avvocatura se collabora con responsabilità con il Ministro ed il Parlamento, siano comunque eque e consentano ai cittadini di poter accedere alla giustizia e ad una difesa di qualità, anche se non hanno grandi possibilità economiche.

che non ne abbiano vantaggio coloro che vogliono ritardare l'esito del processo. Le riforme devono altresì andare nella direzione, sia sul piano del diritto sostanziale sia sul piano del diritto processuale, di dare il più velocemente possibile giustizia a chi dal processo esce come colui che ha ragione. Oggi sempre più cittadini valutano la

Credo che quello che stiamo pagando in termini di sfiducia dei cittadini nello Stato proprio in un settore che, come ho detto prima, è fondamentale, cruciale per la credibilità dello Stato di diritto, sia un prezzo che non possiamo permetterci di pagare oltre, anche perché questo Parlamento ha assunto una decisione estremamente impopolare che è quella dell'indulto. Il Paese pretende che, dopo questa assunzione di responsabilità sull'indulto, si cominci ad amministrare in Italia una giustizia davvero giusta.

ha dichiarato che nel 2006 finalmente si è introdotta un po' di serietà nel dibattito, evidentemente presupponendo che prima non ci fosse. MASTELLA, *ministro ho qui il resoconto stenografico. Oggi ha dichiarato che alcune parti della riforma portata avanti nella scorsa legislatura erano bislacche. Ebbene, lei sa che non sono aduso a porgere l'altra guancia, quindi accetto la sfida proprio su questo piano e farò giudicare non tanto a quest'Aula, che è ovviamente, doverosamente, prevenuta per via degli schieramenti, ma a coloro che in questo momento ci stanno ascoltando nel Paese nel Paese chi è bislacco e chi è serio o poco serio nell'azione per quanto riguarda la giustizia. In primo luogo, credo ci sia stato un equivoco di fondo (lo dico anche ai colleghi che sicuramente sono in buona fede): forse nessuno ha letto il dispositivo della legge che stabilisce appunto questa giornata. questione dice che occorre dibattere non sui servizi resi ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione (cosa che peraltro è estremamente importante), ma sul funzionamento della giustizia e cioè su tutto il coacervo, su tutto il complesso delle azioni che il Ministro della giustizia pone in essere all'interno e all'esterno del Paese. Vorrei partire proprio da questo punto, signor Ministro, dall'attività internazionale, che è estremamente importante. Lei ha partecipato ad un G8, in Russia, perché la presidenza di turno è russa: non ci ha detto neanche una parola su quello che è accaduto al G8, zero; evidentemente l'Italia non ha avuto ruolo in quel consesso. passiamo all'azione europea, che è fondamentale: lei sa benissimo, e dovrebbero saperlo e lo sanno anche i colleghi, quanto sia importante l'azione dei ministri della giustizia in Consiglio GAI.

anche su questo lei non ci ha detto una parola, zero: non sappiamo cosa ha fatto prima, non sappiamo cosa ha intenzione di fare dopo, non sappiamo su quali direttive andrà ad intervenire in Consiglio GAI. Le pare serio tutto ciò, signor Ministro? Io non credo. Le pare bislacco? Io penso di sì: penso che sia veramente bislacco venire qui, in questo consesso, e non dire una parola su temi così importanti e così fondamentali. Infine, la lotta al terrorismo internazionale è un punto che ci ha visti impegnati in prima linea, soprattutto dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Su questo tema noi abbiamo ricevuto moltissime volte attestati di lode dai nostri alleati americani, attestati

forse lei non è al corrente, perché impegnato in questo dibattito, che proprio oggi il procuratore di Milano Minale le ha inviato una lettera

CASTELLI *(LNP)*. Queste sono le due fondamentali questioni affrontate nella sua relazione. Certo, ha affrontato ‑ e questo è un tema importantissimo ‑ la questione dell'eccessiva durata dei procedimenti, ma

perché doveva in qualche modo cercare di riscattare la sua figura e la sua azione di Governo, in questo momento non particolarmente popolari nel Paese - lanciando questo annuncio bomba: i processi dovranno durare cinque anni. Ma lei si è reso conto di cosa significa ciò? Le sottopongo alcuni casi: in una rogatoria internazionale, se i rogati non rispondono, cosa accade? Andiamo ad arrestarli o comminiamo una sanzione al Ministro della giustizia (americano, tedesco o francese) che non risponde alla rogatoria?

Oppure vareremo un'altra legge Pinto, che - come ricordava giustamente il collega D'Ambrosio - è completamente fallita, costa allo Stato centinaia di milioni di euro ed ha ancor di più complicato le questioni? bisogna produrre in Parlamento anche atti concreti, non vaghe promesse. Mi sarebbe piaciuto, allora, signor Ministro, che lei fosse intervenuto su quegli atti concreti - giusti o sbagliati che fossero - che la scorsa legislatura ha visto nascere in Parlamento

qualche provvedimento che, invece, abbiamo messo in campo: ad esempio, la riforma dell'ordinamento giudiziario, talmente vituperata che però poi, alla prova dei fatti, ha dimostrato che su dieci decreti legislativi che abbiamo varato nove vivono

Forse voi non lo sapete nemmeno, colleghi, ma all'interno di questi decreti vi è una riforma fondamentale, che decentra dal punto di vista amministrativo il funzionamento del Ministero della giustizia. È una questione epocale: cosa vogliamo farne? Sono state avviate o meno le procedure? La finanziaria La finanziaria nelle tabelle relative alla giustizia ha lasciato intatti i fondi per tali riforme, che non costavano poco (in totale si trattava di circa 46 milioni di euro all'anno, quindi non una cifra banale); non sappiamo nulla di tutto questo: signor

mi ascolti, senatrice Magistrelli -, lo dice il Governatore della Banca d'Italia, quindi credo una fonte autorevole: «La recente riforma ha favorito una più precoce emersione dallo stato di crisi e una rapida ristrutturazione di imprese, ha snellito e ammodernato le procedure di liquidazione», quindi vede che qualcosa di buono l'abbiamo fatto anche noi? Credo, signor Ministro, che non sia sufficiente

E vengo poi, per finire, se mi lascia un minuto, signor Presidente, all'indulto. Qui bisogna dire una cosa chiara e precisa: il sottosegretario Manconi è venuto a mentire al Parlamento, perché c'è stato un dibattito approfondito sul numero di detenuti che l'indulto avrebbe liberato, ha sempre sostenuto che sarebbero stati liberati 12.000 detenuti, oggi le cifre ufficiali fornite dal suo Ministero ci dicono che a settembre erano 22.000.

di accettare le dovute conseguenze su questo tema e di prendere provvedimenti nei confronti di un Sottosegretario che è venuto scientemente a mentire. Infine, ha dichiarato: ha dichiarato: «Voglio anche dire con forza che la stella polare della mia azione di Governo non sono associazioni o gruppi professionali, pur autorevoli e influenti, bensì i cittadini». Quindi, lei ci dice che l'indulto lo ha deciso a favore dei cittadini. Io la sfido: venga fuori con me alla fine di questo dibattito, noi l'abbiamo vista brindare con i detenuti quando l'indulto è stato approvato,

parlerò molto meno dei 18 minuti a mia disposizione, voglio tranquillizzare i colleghi presenti. Sono l'unico del Gruppo UDC che interviene, perché faccio parte della Commissione giustizia, ma dico in premessa che non sarà un intervento di tecnica giurisdizionale; nell'Aula del Senato ho l'impressione che si debba discutere di una questione che precede qualunque discussione tecnica, ovviamente le discussioni tecniche le vedremo man mano che il Governo presenterà i disegni di legge ai quali ha fatto riferimento il Ministro, ma qui vi è una questione che premette le questioni tecniche, che viene prima e che non è stata oggetto di nessuna dichiarazione da parte del Ministro. Vorrei che su questo punto si capisse perché vi è stato questo silenzio. Signor Ministro, io mi limito soltanto ad informarla di un fatto che attiene ad un caso clamoroso di malagiustizia, ve ne sono tanti, ma ce n'é uno clamoroso che ha un valore politico enorme: il 10 gennaio scorso, cioè pochi giorni fa, il tribunale di Latina ha assolto, su conforme richiesta del pubblico ministero del tribunale, il senatore Michele Forte da gigantesche e spaventose accuse, che avevano portato persino all'arresto in carcere del senatore Forte, perché il fatto non sussiste, tredici anni dopo l'arresto, signor Ministro. Quell'arresto non è avvenuto per caso, un giorno qualunque, ma è avvenuto nel marzo del 1993 e vorrei ricordare al signor Ministro che eravamo nel pieno di quella vicenda che qualcuno di noi ha ritenuto costituisse una sorta di colpo di Stato: arresti a ripetizione di esponenti politici locali e nazionali del partito democristiano e di partiti alleati della Democrazia Cristiana, che si sono tradotti non solo in normali assoluzioni, sulla base dell'affermazione che il fatto non costituisca reato o di non averlo commesso, ma qui siamo in presenza del fatto clamorosissimo che tredici anni dopo si dice che il fatto non sussiste. sussiste. Non chiedo provvedimenti giudiziari nei confronti di chi all'epoca ha chiesto l'arresto, né di chi lo ha deciso, ma mi chiedo: una cosa del genere non pone anche a lei la domanda di cosa sia successo allora? E se non rispondiamo a quella domanda, come facciamo ad affrontare i problemi dell'ordinamento giudiziario del nostro Paese, per così dire, come se si trattasse di normali vicende giurisdizionali? Lo dico perché alcuni dei colleghi oggi qui presenti sono stati illustri esponenti delle procure della Repubblica hanno adottato quei provvedimenti, non so se per conseguenza di ciò che è avvenuto allora, ma certamente in conseguenza del fatto che allora sono stati fatti scomparire "interi" esponenti del potere politico. Perciò la domanda è se

avvenuti in tante parti d'Italia a danno delle stesse persone ed esponenti dei medesimi partiti politici, oppure di fatti straordinari. Rispetto al suddetto problema l'attuale Governo che intenzioni ha? Il Governo di centro-sinistra dice qualcosa o non dice nulla

a cercare la più larga intesa sulle questioni giudiziarie, nella convinzione che vicende del genere non possono essere vissute in termini di vendetta e di contro vendetta, è interessato a sapere se esiste una politica giurisdizionale in questo Paese, di cui il Governo attraverso il Ministro è espressione, in ordine a questo problema fondamentale. Se esiste, noi vorremmo sapere qual è.

che si possa affermare soltanto una sorta di principio in base al quale da un lato vi sono le leggi vergogna e dall'altro le leggi oneste. Siamo stati in presenza di un fatto di straordinario rilievo politico e costituzionale sul quale abbiamo il dovere di sapere se esiste o no

di qualunque questione giurisdizionale. Ho voluto citare non un generico caso di un condannato democristiano, ma di chi dopo 13 anni viene assolto perché il fatto non sussiste. Ancora una volta mi chiedo come potesse essere ritenuto sussistente un fatto all'epoca del 1993 nei confronti di un sindaco di una grande città della provincia di Latina, se non per il fatto dell'appartenenza di questa persona ad un partito politico. Se così è, mi chiedo cosa sia successo allora. È interessata questa maggioranza a sapere cosa sia accaduto allora o no? I colleghi dell'opposizione, che all'epoca hanno concorso ad affermare il principio della normalità di un intervento giurisdizionale a danno degli esponenti dei partiti di Governo dell'epoca, hanno anche loro il diritto di chiedere cosa sia successo allora o no? Vogliamo fare chiarezza su un fatto che ha rappresentato l'origine della situazione politica italiana dal 1994 in poi? Sono molto lieto che sia presente il collega Follini ad ascoltare queste considerazioni perché è stato segretario dell'UDC fino a qualche tempo fa:

che siamo in presenza di due questioni di straordinario rilievo politico, politico l'uno - le leggi elettorali - politico l'altro, il rapporto magistratura-potere politico? Tali due questioni, signor Ministro, sono a premessa del suo intervento. Per questo non siamo in grado di esprimere un'opinione sulla sua comunicazione,

A noi interessa ancora una volta sapere se in premessa questa maggioranza politica è consapevole del fatto che vi sono due questioni politiche all'origine di questa vicenda dal 1994 in poi in Italia, senza dare risposta alle quali non vi è possibilità di affrontare né la legge elettorale né i problemi specifici dell'ordinamento giudiziario. Per queste ragioni, senatori, signor Ministro, non possiamo esprimere un parere favorevole alla sua relazione; non presentiamo una nostra mozione in tal senso ma continuiamo a chiedere che lei risponda, anche da questo punto di vista, alla questione fondamentale: la premessa dell'ordinamento giudiziario. Fino a quel momento non saremo in grado di dare un'opinione. *(Applausi

colleghi senatori, il dibattito sarebbe stato utile se il Ministro, invece di attardarsi in un catalogo di generiche intenzioni, alcune buone altre palesemente errate nel fondamento, avesse dato a noi la possibilità di una interlocuzione più precisa. Se il dibattito deve servire ad assolvere a una funzione autoconsolatoria per una periodica esercitazione ministeriale, ben venga il dibattito! Se, invece, esso deve servire a focalizzare i temi della giustizia, in un momento particolarmente delicato della vita del Paese, il Ministro, secondo il nostro apprezzamento, non ha dato un grande contributo. Sarebbe stato molto più utile che il Ministro avesse fornito non l'anticipazione epigrafica dei suoi disegni di legge, ma il testo di questi disegni di legge per metterci in condizione di poterli subito valutare. Oggi ci troviamo di fronte ad una rappresentazione che non ci convince, che ci pone in una situazione di grande criticità e che, comunque, permette a noi di Alleanza Nazionale di offrire sul tema della giustizia, al di là dei luoghi comuni e delle ovvietà, un contributo su temi particolarmente interessanti e importanti. Parlare della giustizia come di una necessità del Paese è cosa ovvia e pacifica. Parlare della giustizia come del crocevia o dello snodo istituzionale più delicato in questo momento significa riaffermare una definizione che da almeno 15 anni si trascina. Abbiamo bisogno invece di andare a fondo e di capire sino in fondo, al di là della eleganza formale con cui si esprime il Ministro e al di là delle distanze che prende, sia nei confronti della classe forense, ma minori distanze assume nei confronti della classe magistratuale,

ma, proprio sul tema dell'indulto devo oggi farle una critica precisa. Non vi è stato alcun apprezzamento di condizioni atte a far sì che coloro che uscivano dalle carceri potessero trovare situazioni non dico di accoglienza ma di pari normalità, che avrebbero impedito il loro immediato rientro negli Non sono convinto che oggi nelle carceri italiane, come ella si esprime, vi siano le migliori condizioni di umanità. L'informatizzazione della cartella clinica del detenuto è una buona aspirazione, ma chi frequenta professionalmente le carceri sa che oggi le condizioni di promiscuità, la mancanza di lavoro e la carenza di adeguati servizi igienici, infermieristici e medici sono una costante connotazione negativa su quasi tutto il territorio nazionale. Ecco perché il suo ottimismo in materia non lo possiamo condividere. Quando lei parla del *gap* che ancora divide nel settore civile le cause di nuova iscrizione da quelle definite fa riferimento ad una realtà che negli ultimi anni è andata migliorando. Ma quando da queste affermazioni di principio scende sul terreno pratico delle proposte queste si mantengono su un'astrattezza così aerea da rasentare l'impossibilità del colloquio e dell'interlocuzione.

di costi, di spreco di risorse e di ottimizzazione di energie materiali e intellettuali nel Paese avesse proposto il recupero di queste ultime attraverso una modificazione del reticolo giudiziario. Si faccia promotore della revisione delle circoscrizioni giudiziarie se ne ha il coraggio, signor Ministro. La maggiore sacca di inerzie e letargie sul piano dei costi è nell'irrazionale distribuzione del reticolo giudiziario. Ma non c'è coraggio nell'affrontare questi problemi. Sono problemi che riguardano la struttura ordinamentale. Sono problemi che riguardano lo *chassis* su cui deve camminare la giustizia nel nostro Paese. Qui veramente ci vorrebbe un'inchiesta *bipartisan* fra tutte le parti politiche per rendersi conto che non è possibile tenere in piedi un'impalcatura che geneticamente si riallaccia ad anni che risalgono al sorgere dell'Unità d'Italia, addirittura a prima del 1860, signor Presidente. Mi sarei aspettato che sul piano delle riforme ordinamentali, invece di sciorinarci il solito rosario di ovvietà in ordine alla valutazione di professionalità, ci fosse stato detto vuole modificare i consigli giudiziari stabilendo la presenza decisiva, cioè con diritto di voto, degli avvocati e delle componenti sociali dei Comuni e delle Regioni che insistono nei distretti. non ci ha detto nulla. Ci ha parlato di una valutazione di professionalità che, come ha ricordato il senatore Palma, appartiene a una delle peggiori e deteriori prassi corporative della magistratura:

delle riforme ordinamentali, ella avesse posto il problema delle carriere non attraverso la ripartizione della distinzione delle funzioni su base distrettuale: soltanto chi conosce la storia dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario sa che il passaggio da requirente a giudicante scivola come un bicchiere d'acqua, senza alcuna valutazione intrinseca e seria. e seria. Se vogliamo andare verso il processo di parti, dobbiamo avere il coraggio di affrontare il problema della separazione delle carriere una volta per tutte. Prima era considerato un tema soltanto di una parte dell'avvocatura, ma su di esso si misurano i diritti civili dei cittadini in un Paese normale. Mi sarei augurato, signor Ministro, che ella avesse affrontato, sul piano della riforma ordinamentale, un altro tema: la vogliamo finire con la giustizia corporativa dei magistrati e - dico anch'io - degli avvocati? dell'articolo 111 della Costituzione, la terzietà del procedimento riguarda anche il procedimento disciplinare. Perché la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura deve avere al suo interno una maggioranza preponderante di magistrati? Perché gli avvocati devono essere giudicati soltanto dagli avvocati? Non sono cittadini come gli altri? Se vogliono essere cittadini intrinseci ai destini del nostro Paese, devono accettare il principio non solo dell'imparzialità, ma della visione terza del giudice. Questo è il coraggio che noi le richiedevamo, perché va nella direzione di una democrazia compiuta sul piano della giustizia. Ho apprezzato le sue affermazioni di principio in ordine alla volontà di ridurre i tempi del processo

Vogliamo imporre termini perentori alla definizione dei processi? Sono affermazioni di carattere ideologico-politico. Se lei pensa effettivamente di poter ridurre gli anni del processo a cinque,

In Italia, nel Paese della disquisizione dialettica, del capello spaccato in due, prevediamo termini vincolanti allo svolgimento del processo? È un'affermazione di puro principio che non serve a nulla, perché priva di qualsiasi contenuto.

ma non vorrei che quei dati si riferissero anche alle questioni di giurisdizione, materia diversa dalla competenza. Per concludere, signor Ministro, le debbo dire sinceramente

Questa collettiva e collegiale udienza di programmazione con i cancellieri, gli avvocati e i giudici non servirà a nulla. Sarà un altro segmento di intoppo nello svolgimento fisiologico del processo. Ecco perché, signor Ministro, questi sono pannicelli caldi.

Così come non è possibile ipotizzare che si possa prevedere un patteggiamento per coloro che possono usufruire dell'indulto. Ma chi può usufruire dell'indulto non patteggia: attende che la giustizia faccia il suo corso eterno. Non vi è alcun interesse, né alcuno stimolo a patteggiare. E ancora, signor Ministro, mi sarei aspettato qualche parola in più su un tema scottante e molto importante che dovrebbe interessarla, visto che lei è campano e dunque appartiene ad una delle Regioni segnate dalla criminalità organizzata, dall'occupazione del territorio da parte della mafia, dal crescere e irrobustirsi dell'antistato.

invece al totale fallimento in tutta Italia della gestione dei beni confiscati. Perché non ipotizzare un'agenzia speciale? Sottraiamo all'Agenzia del demanio competenze che non è stata in grado di mettere in moto, ricreiamo meccanismi virtuosi perché

Lei ha fatto riferimento alle intercettazioni e poi al patteggiamento. Sono passaggi del tutto secondari. Il patteggiamento in appello è molto ben praticato e serve a deflazionare in appello le spese per le intercettazioni che andrebbero riviste in maniera adeguata. è una obbrobrietà giuridica che debbo denunciare qui in Senato. Lei vuole stabilire una prescrizione prima che si formi il giudicato penale andando a cozzare contro tutti i princìpi giuridici che hanno retto la storia del diritto nel nostro Paese. Come si fa a stabilire la prescrizione di un reato prima che si sia consumato e sia arrivato a definizione? Non credo che con questa sua - forse nelle intenzioni - provocatoria relazione possa innescarsi un dibattito serio. Noi abbiamo cercato di apportare il nostro contributo. Ci auguriamo di poter leggere i suoi disegni di legge, ma oggi mi vedo costretto a dire, ripetendo una frase che appassionò negli anni Settanta un noto politico italiano: purtroppo lei si è espresso *nisi caute, nisi caste*.

Come apprezzo molto la posizione da lei assunta, signor Ministro, rispetto all'ipotesi dell'abbassamento dell'età punibile. La ringrazio sia personalmente che a nome del mio Gruppo Vorrei, tuttavia, porre l'accento e richiamare ulteriormente la sua attenzione sulla questione delle politiche penitenziarie di fondamentale importanza per la ripresa del rapporto di credibilità tra cittadini ed istituzioni. Come lei, signor Ministro, ha ricordato nella sua relazione, non è soltanto la politica ad essere suscettibile di giudizio negativo da parte dei cittadini ma l'intero sistema giudiziario che produce elementi di sfiducia, insofferenza e incomprensione nelle persone. Questo stato di cose si è con più forza manifestato con l'approvazione del provvedimento - per me sacrosanto - dell'indulto che ha generato, a causa di una relazione verso l'esterno viziata nella forma e nella sostanza, disorientamento diffuso in merito alla certezza della pena e alla tutela della legalità. Il tutto, probabilmente, anche a carico di molti tra noi che, pur avendolo votato, lo hanno poi rimesso in discussione, testimoniando un sistema che spesso, purtroppo, si disconosce a scapito della credibilità non solo della politica nel suo rapporto stretto con le istituzioni ma, cosa ancora più grave, della dignità e dell'autenticità dell'attività legislativa del Parlamento stesso. I principali problemi delle carceri italiane riguardano, in particolar modo, l'assoluta inadeguatezza delle strutture prive dei necessari servizi, caratterizzate da un tale sovraffollamento che anche i detenuti che dovrebbero essere assegnati a celle singole per ragioni di giustizia, disciplinari o cautelari - ad esempio i detenuti in regime di EIVC sono costretti a vivere con altri detenuti. Gravissima è anche la condizione strutturale strettamente carente che penalizza l'assistenza sanitaria in carcere. Abbiamo inoltre rilevato, in base ad ispezioni effettuate in alcune carceri e anche dalle dichiarazioni di molti detenuti che ci scrivono ogni giorno, l'inerzia e l'atteggiamento poco collaborativo dell'ufficio trasferimenti del Infatti, molte istanze di trasferimento dei detenuti, basate su ragioni di studio o di avvicinamento al nucleo familiare, vengono sistematicamente rigettate, e spesso, purtroppo, violando il diritto allo studio, all'istruzione e alla formazione culturale, tutelati peraltro dagli articoli 33 e 34 della nostra Costituzione, e anche in violazione del principio di territorialità della pena che garantisce al detenuto la tutela dei rapporti familiari. Il diniego delle istanze di trasferimento è assoluto poi per i detenuti in regime di EIVC per i detenuti in regime di EIVC o AS, perché la loro detenzione è prevista in istituti lontani dai familiari e comporta l'impossibilità di richiedere trasferimenti per motivi di studio, nonché l'impossibilità di partecipare a programmi previsti solo per detenuti comuni. Rispetto a tali problematiche l'impegno del nostro Gruppo è stato particolarmente intenso e si è svolto non soltanto mediante la presentazione di atti di sindacato ispettivo, ma anche con la presentazione di alcuni disegni di legge, tra i quali l'Atto Senato n. 1230, in materia di diritto di reclamo dei detenuti e degli internati, e l'Atto Senato n. 1191, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti. Tali disegni di legge mirano a garantire una più ampia tutela giurisdizionale ai detenuti riguardo agli atti della amministrazione penitenziaria lesiva dei loro diritti. Infatti, la normativa sull'ordinamento penitenziario, come attualmente regolata della legge n. 354 del 1975, prevede una disciplina fortemente restrittiva nel merito. Dobbiamo ricordare, onorevoli colleghi, quanto sancisce l'articolo 64 delle regole penitenziarie europee: la pena detentiva non deve aggravare le sofferenze inerenti a essa, con espresso riferimento alla sofferenza data dalla privazione della libertà personale e alla limitazione della libertà di movimento. Del resto, i diritti alla salute, alle relazioni affettive, alla riservatezza della corrispondenza, alla *privacy*, alla dignità, alla partecipazione al percorso trattamentale non sono e non possono essere suscettibili di atteggiamenti discrezionali e arbitrari perché non è su tale limitazione che deve fondarsi la pena. Al contrario, la tutela di tali diritti rafforza la funzione rieducativa e la finalità del reinserimento sociale della sanzione penale stessa. Ad evitare un eccessivo incremento del carico giudiziario per la magistratura di sorveglianza si è previsto, con un ulteriore disegno di legge del nostro Gruppo parlamentare, l'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, che svolga un ruolo qualificato preventivo, mediatorio e propositivo rispetto alle legittime richieste dei detenuti, alleggerendo in tale modo anche l'attività del giudice. Infine, per ridurre l'effetto dell'incarcerazione di massa prodotta dalla legge *ex* Cirielli, il nostro Gruppo parlamentare ha presentato un disegno di legge di riforma degli istituti della recidiva e della prescrizione, tale da eliminare le restrizioni, poste dalle legge n. 251 del 2500, all'accesso ai benefici penitenziari nei confronti dei recidivi. Auspichiamo qui un forte sostegno suo, signor Ministro, e anche dei nostri onorevoli colleghi a tali proposte legislative che mirano, in conclusione, a garantire la funzione rieducativa della pena

Signor Presidente, ho apprezzato particolarmente la relazione svolta dal ministro Mastella per due aspetti che potremmo definire macropolitici che, pur non affrontando tematiche politiche specifiche, offrono però delle indicazioni di direzione di sistema complessivo che io considero importantissime. è politico-metodologico e recupera un approccio di sistema molto caro al Presidente della Repubblica. Le riforme importanti che affrontano i problemi del Paese - e quello della giustizia è un signor problema - non si fanno contro qualcosa o contro qualcuno, ma per modernizzare la società. Ecco perché devono essere fatte insieme, devono tendenzialmente essere condivise, discutendo serenamente il merito ed affrontando consapevolmente i problemi, senza soluzioni preconcette o precostituite, forgiate sulla scorta di valutazioni ideologiche o, peggio, di schieramento; non improntate signor Ministro a puerili rivincite o ad ingenerose smanie di controriforma. Su questo tema il Ministro - nell'augurarsi che il metodo del confronto libero e della partecipazione concreta prevalga su quello del muro contro muro che, quasi sempre, era stato utilizzato nella scorsa legislatura parlando della rivisitazione della riforma dell'ordinamento giudiziario, ha testualmente dichiarato: «L'intervento del Parlamento ha rappresentato, a mio avviso, un atto di grande responsabilità che se, da un lato, ha realizzato un'utile sintesi, seppur non perfetta, sostenuta da un largo consenso politico (più al Senato di quanto si è verificato alla Camera), dall'altro rende ora necessaria un'ulteriore, urgente iniziativa legislativa». Ha poi comunicato all'Aula, nella precisazione fatta qui in Senato, che il provvedimento relativo a quella parte di riforma sospesa è stato depositato al Consiglio dei ministri. Ma il ministro Mastella sa bene che quell'atto di grande responsabilità che ha determinato una rivisitazione, in buona parte condivisa da maggioranza ed opposizione, della riforma, è stato possibile per il suo grande coraggio e per la tenace determinazione di alcuni senatori - a partire da chi vi parla e continuando, tra gli altri, i colleghi Salvi, Centaro, Caruso e Castelli - che hanno nell'occasione (mi riferisco a quella parte di riforma dell'ordinamento giudiziario che non è stata sospesa e che è riuscita invece ad essere rivista, perfezionata ed approvata definitivamente) cercato di comprendere che «la centralità del sistema giustizia, architrave dell'ordinamento democratico per la difesa dei diritti individuali e la sicurezza dei cittadini, straordinariamente importante per la competitività economica del nostro Paese, costituisce» - come appunto dice il Ministro - «una priorità assoluta che deve far sentire tutti consapevolmente vincolati ad un metodo di confronto pacato ed aperto». Ma lei comprende bene, signor Ministro, che questo approccio non sarà sempre né facile né agevole, anzi sappiamo che molto spesso si tenderà a far prevalere ancora una volta quella politica del muro contro muro che non solo non è consigliabile data l'importanza della posta in palio, ma onestamente non è nemmeno praticabile in un'Aula come quella del Senato che ha invece bisogno di quella tenacia e di quel coraggio che ha dimostrato già in altre occasioni. La seconda considerazione che lei ha svolto, signor Ministro, e che considero straordinariamente importante è quella di voler considerare al centro di questo percorso riformatore un unico fondamentale soggetto: il cittadino, l'utente. In buona sostanza, ci ha ribadito che le riforme non vanno fatte per le singole associazioni di categoria, ma per la gente comune che deve poter fruire con tranquillità del servizio giustizia, superando una prognosi di inaffidabilità del sistema che oggi è generalmente prevalente. Anche questo proposito, alto e nobile, sarà difficile da realizzare perché, durante il percorso, non saranno poche le spinte ed i tentativi corporativi di condizionamento. Ma, se manterrà salda la rotta e non smarrirà la stella polare di riferimento, anche questa difficile missione - che lei ha definito essere, in parte, una missione impossibile, secondo le affermazioni raccolte ieri alla Camera dei deputati - potrà essere realizzata e, sempre se si atterrà a quella stella polare, ci troverà al suo fianco. Sul punto, però, mi permetto di aggiungere che la tutela dei diritti, la difesa delle ragioni e la sconfitta delle ingiustizie, i cittadini possono realizzarle - all'interno del sistema giustizia - soltanto recuperando all'alta professione forense, al ruolo dell'avvocato, una dignità che molto spesso è dimenticata. Dignità che, quasi sempre, è del cittadino prima che del difensore. Se, come detto, non possono che condividersi l'approccio ed il metodo che motivano ed animano il progetto di riforma illustrato, che resta però lo voglio dire anche al collega Peterlini che è un po' distratto - un progetto tendenziale e di massima, certamente non esecutivo, sembra necessario soffermarsi - mi consentirà signor Ministro - con atteggiamento critico-costruttivo su alcune delle intenzioni riformatrici indicate, premettendo che tutte le idee progettuali - chiaramente da specificare - avranno bisogno di essere corredate delle necessarie risorse straordinarie, certamente necessarie per riconvertire una macchina giudiziaria che oggi, per onesta ammissione dello stesso Ministro guardasigilli, si presenta inaffidabile, improduttiva ed inefficace. Nell'Aula del Senato lei ci ha parlato della California, dei ricercatori, immaginando di poter coniare un modello che potremmo definire del *California dreaming*, ricordando un poco la nostra infanzia. Non so se sarà un modello applicabile, ma è una scommessa che in qualche modo sentiamo di voler fare: recuperare prima il progetto e poi fare in modo di reperire le risorse. L'accelerazione dei processi, vera e propria questione nazionale in termini di garanzie individuali, competitività del sistema economico e prestigio internazionale del nostro Paese, ed obiettivo principe della riforma, si potrebbe risolvere - lei lo ha detto - prefissando una durata massima complessiva di cinque anni per i tre gradi di giudizio, tanto per i processi civili, quanto per quelli penali, sperimentando una formula temporale che potremmo chiamare

atteso che il numero dei processi - civili e penali - aumenta, come lei ha detto, in misura esponenziale ed i dati relativi alle giacenze medie palesano situazioni allarmanti: per i processi civili in fase di appello si registra una giacenza media pari a 44 mesi (oltre 3 anni e mezzo, quindi quasi il doppio di quanto lei prevede nella formula), mentre per il primo grado abbiamo una forbice di giacenza che va dai 3

che, all'interno di un percorso nel quale, attualmente, alcuni rinvii di udienza purtroppo superano gli ipotizzati limiti di fase, alcuni aspetti suscitano

Quanto al processo civile, signor Ministro, avverto l'obbligo di precisare che, all'interno di un percorso nel quale, attualmente, alcuni rinvii di udienza purtroppo superano gli ipotizzati limiti di fase, alcuni aspetti suscitano forti perplessità, l'intento di condizionare l'esito della domanda giudiziale con l'istituzione di sanzioni processuali a carico della parte che abbia, senza giustificati motivi (come diceva il collega Buccico con cui sono d'accordo), rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla controparte o dal giudice; la trasformazione dell'appello, oggi mezzo di impugnazione con potenziali effetti devolutivi, in sostanziale ulteriore giudizio di terzo grado, prevedendosi la possibilità di proporlo solo per motivi chiusi e specifici; la razionalizzazione dei meccanismi di liquidazione delle spese processuali, mediante la previsione di incentivi per l'ipotesi di minor durata del processo. Quanto agli interventi sul processo penale, per il quale pure

al tempo necessario per fissare l'udienza preliminare ed arrivare al giudizio di primo grado, molto spesso nel processo penale si giunge oltre il limite di fase che lei prevede. Rispetto al processo, *prima facie*, mi permetto di dire che non ci è dato comprendere i limiti della ipotizzata proposta di revisione del regime delle nullità, con l'introduzione di più rigide preclusioni temporali, così come appare allo stato incomprensibile l'asserita logica riequilibratrice alla base del radicale intervento in materia di prescrizione, che si intende fissare ad un momento anteriore alla formazione del giudicato parziale. La parità delle parti processuali, nell'ottica del Ministero di via Arenula, imporrebbe che, come da un lato al pubblico ministero è preclusa l'impugnazione della sentenza di assoluzione, così l'eventuale sentenza di condanna in primo grado dovrebbe comportare la preclusione di ogni prescrizione per l'imputato.

giacché da sempre risponde esclusivamente alla logica del disinteresse dello Stato alla punizione in ragione del tempo trascorso dalla presunta commissione del reato. Parimenti incomprensibile allo stato appare la logica del *do ut des,* che ispira l'introduzione di ulteriori limiti temporali per il patteggiamento. Conclusivamente, lo spirito e le intenzioni della sua relazione sono da condividere; mi permetto soltanto di dire che il cittadino deve rimanere, come lei afferma, al centro del percorso riformatore e al cittadino interessano certamente i tempi ragionevoli e certi, ma all'interno di un percorso processuale nel quale il sistema di garanzie non possa essere mai scalfito o depauperato da alcuno. *(Applausi

Leggo dai dispacci di agenzia: «I giudici della Consulta hanno dichiarato illegittimo l'articolo 1 della legge, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello contro la sentenza di proscioglimento. illegittimo anche l'articolo 10, nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima del 9 marzo 2006, quando è entrata in vigore la legge Pecorella». Questo, per ragioni solo di natura formale e per dire, in relazione ai rilievi che sono fatti a me che, come ho detto, ognuno ottiene rilievo a rilievo; quindi, io accetto la mia parte, vedo che invece il Parlamento ha avuto i rilievi da parte della Corte costituzionale.

devo chiedere alla mia maggioranza, al mio Governo (e spero anche nel consenso dell'opposizione), quali sono i cardini su cui si esce dall'emergenza del problema giustizia e si ritiene di risolvere tale angoscioso problema. Questo mi pare evidente.

lasciamo stare le cose come stanno. Io debbo dire la verità: sarà perché ragiono come uno che è arrivato a valutare questo mondo, quindi vedendo gli apporti di grande intelligenza di tanti magistrati ed avvocati, ma vedendone anche i limiti, per me nel complesso la giustizia non funziona.

Non ho nulla da tenere in serbo che non possa recare come mia opinione e come frutto dell'opinione del Governo in sede internazionale, così come non saggiare i contributi provenienti in futuro anche da questo punto di vista da parte delle opposizioni. È vero oppure no che da anni in maniera inquietante (come cittadino provo una forma di pudore

Tutti siamo chiamati, perché cinque anni fa e pochi mesi fa c'eravate voi, oggi ci siamo noi. Non voglio ascrivere a me il merito di quello che, eventualmente, si fa; voglio che sia merito del Parlamento come tale,

tranne che non sia una sorta di strano mostro (che riesce a concepire, come padre e madre assieme e contemporaneamente, questa idea dell'indulto che si è verificata). A mio parere,

meglio della Camera. Siamo arrivati ad un comportamento e ad uno stile privi di pregiudizio: vi era il giudizio. Abbiamo orientamenti diversi, questo mi pare evidente; credo, però, che, al di là di essi, sappiamo tutti che il cittadino che riflette su questo stato d'insufficienza e di incapacità della giustizia chiede a tutti, qua dentro, di fare qualcosa.

non si è ancora opacizzata la mia grande passione per vivere questo momento con l'intensità necessaria, che porta con sé il dovere etico di far qualcosa in risposta. Da questo punto di vista, infatti, non voglio che siano ingaggiate

rilievi e sconnessioni che vengono quotidianamente emergendo nel rapporto tra cittadino e disfunzione dal punto di vista giudiziario. Cinque anni, il tratto investigativo, eccetera: la cosa singolare - voglio

che la pacca che si può dare amabilmente ad una ragazza una volta si segnala come pena e come reato, un'altra volta invece come fatto goliardico; ma è possibile che sul piano del giudizio bisogni arrivare in Cassazione? Questa è la verità, questo è quanto rivelano le cronache. Allora, non sono così distante né così fuori dal mondo: segnalo soltanto elementi ontologicamente presenti alla storia corrente, alla quotidianità dei cittadini italiani. Ecco perché

un'eccezionalità in ordine al problema della giustizia, occorre anche accampare poste di bilancio che siano molto più eclatanti di quelle registrate quest'anno. Sarebbe sciocco, da parte mia, un'ipoteca e dire al Paese che per quest'anno sarà così, però diciamo la verità: a chi mi chiede quando arrivano queste proposte di riforma, debbo anche dire che il Parlamento in realtà a volte non è in grado di smaltire quello che arriva;

nonostante i disegni di legge vengano approntati; e da questo punto di vista mi pare che i rilievi che emergono dal senatore Maccanico, che ha fatto proposte al riguardo, non siano eccedenti o esorbitanti o eccessivi, ma siano molto ragionevoli e comprensivi di queste ragioni. È ovvio che l'ipoteca che si pone è un'ipoteca - voglio dirlo per cinque anni. Cioè, questo è un programma che vale per cinque anni, le proposte che faccio non valgono di qua a tre mesi, valgono nello spazio concesso dalla mia attività, mi muovo nel cono d'ombra di questa maggioranza, se questa maggioranza regge per cinque anni, altrimenti sarà per chi sarà.

com'è capitato oggi, dovendo contenere i conti, ma sia un Paese che vada in avanti, si riprenda e faccia paracadute rispetto al declino e ci siano le risorse necessarie anche e soprattutto nel settore della giustizia. Questa è la mia ambizione, questa è la modesta rincorsa di un operatore politico, queste sono le ragionevoli proposte che mi sono permesso di sottoporre alla vostra attenzione. Poi, quella che sarà la figurazione, gli elementi giuridici di quelle che sono sono inflessioni del mio dialetto giuridico esposto a voi li tradurremo in italiano più corretto giuridicamente - che volete che vi dica? - però mi pare che le impazienze dell'opinione pubblica siano su un tono e su un'altezza tale che richiedano a tutti quanti noi una risposta celere, certa, non esuberante, ma manifestamente accertata rispetto a quello che è il dato dell'oggettività con cui ci si ritrova a dover fare i conti in ogni circostanza.

che si può lavorare anche per richiedere interventi massicci da destinare come risorse al settore della giustizia. In alcuni casi sono risorse aggiuntive, in altri sono fondamentali. Ricordo, in

tale risoluzione non per disciplina di partito ma per convinzione, perché riteniamo che il Ministro abbia fatto bene a chiedere un contributo al Parlamento. Riteniamo che l'approccio al problema sia quello giusto, cioè

di alcune leggi, le cosiddette leggi vergogna (le abbiamo definite noi così) o al mantenimento fermo del principio dell'inseparabilità delle carriere; una serie di posizioni che ci trovano d'accordo e rispetto alle quali

Crediamo che serva a mettere il Ministro in una posizione, in cui probabilmente già si trova, di totale sintonia con il programma dell'Unione su questi temi e, ove mai fosse necessario, probabilmente serve a raddrizzare la

cento dei magistrati possa essere destinato all'80 per cento di questi processi, che per una legge da noi non voluta finiranno con l'essere abbastanza inutili, cento continui a lavorare su processi che invece avranno uno sbocco finale di condanna o di assoluzione. È un esempio, serve per dire che lo spirito con il quale abbiamo lavorato a tali proposte è quello che lei, signor Ministro, invocava: uno spirito di leale collaborazione tra forze politiche della stessa coalizione, che probabilmente possono anche registrare sensibilità diverse su alcune questioni, ma che sanno che solo la sintesi feconda

colleghi senatori, oggi ci siamo ritrovati a dibattere sulla questione giustizia, tema essenziale per una Nazione che punta sullo Stato di diritto, Stato di diritto già preannunciato al tempo del provvedimento di indulto. Reputo opportuno procedere con un resoconto che non sia semplice e sterile elencazione, bensì quadro sintetico e significativo dello stato dei fatti, perché solo con dati alla mano si può procedere tracciando linee programmatiche efficaci. Infatti, si disse allora e si è mantenuto adesso che l'indulto non era espediente isolato, ma strategia mirata, *incipit* per una riorganizzazione onnicomprensiva e, per quanto epocale, solo un passaggio. Si imponeva un intervento senza indugi per ripristinare legalità ed efficienza e, contro ogni critica, parlano i fatti. Si è registrato un sensibile calo dei reati che, ovviamente, giova a tutti, contrariamente a quanto si vuole far apparire. Ciò nonostante, colleghi senatori, non possiamo fermarci, nascondendoci dietro false verità. Di fatto, condivido con il Guardasigilli il forte rammarico nel constatare, a malincuore, che si diffonde tra la gente un senso di insoddisfazione nei confronti della giustizia. Se i cittadini sono sfiduciati o addirittura - come ha riferito il ministro Mastella - si sentono impotenti, le istituzioni hanno l'obbligo di intervenire. Il piano d'intervento del Guardasigilli è un miracolo? Certamente no, ma ci stiamo attrezzando per far funzionare una macchina che dev'essere perfetta e dare garanzie a tutti i cittadini. È ovvio che si deve combattere questa generale crisi di affidabilità, intervenendo sulle lungaggini pericolose e deleterie ed accelerando i tempi di analisi di tutti quei provvedimenti relativi all'amministrazione giudiziaria. Il passo decisivo è sicuramente abbreviare la strada della giustizia, cioè ridurre i cosiddetti tempi di giacenza e di durata dei processi. Chi, dinanzi all'odierna prospettiva di durata di una causa, non si sentirebbe atterrito, sfiduciato e perfino demotivato al punto di non procedervi affatto? Orbene, in tal senso va il giusto monito del Ministro a contenere nei cinque anni il giudizio. E per non alimentare la disaffezione del cittadino alla giustizia, occorre intervenire su udienze di programmazione che scandiscano tempi e modi del processo sia civile che penale, sull'esaltazione del potere di conciliazione del giudice, sulla confermata intenzione di ammodernare i processi, modificando i tempi di prescrizione e le questioni di nullità e competenza. Comunque, senza soffermarmi oltre sui particolari del piano di riforma e mantenendo sempre aperta la porta a possibili e sostenibili integrazioni, vorrei estrapolare qualche altro dato fondamentale, degno di essere menzionato: ad esempio, l'opportuno intervento sulla preparazione di chi è chiamato a giudicare. La carriera è e deve restare unica, ma cadenzata da scelte e controlli della professionalità acquisita. Cari colleghi, se vi domandassi se vi domandassi retoricamente a quale medico affidereste le cure per la vostra persona è ovvio che, potendo scegliere, tutti optereste per lo specialista che si è tenuto costantemente aggiornato, superando magari periodiche valutazioni, cioè quello più competente: lo stesso dicasi per la giustizia. È per questo motivo che il ministro Mastella parla di uomini giusti al posto giusto, di magistrati istruiti attraverso sistemi di selezione efficaci che consentano di attribuire gli incarichi direttivi solo a professionisti validamente formati. Lo ripeto: il piano di riforma non è un miracolo, ma un tentativo di consolidare tra politica e magistratura il clima di serenità ultimamente ritrovato, che superi la fase delle interferenz*e tout court* e si arricchisca nel confronto. Bisogna mantenere la giusta autonomia tra i due poteri; è un equilibrio molto difficile. Concludendo, intendo ribadire che tutti i temi di matrice giudiziaria meritano una riflessione parlamentare profonda che dia spazio e voce alle categorie interessate ed abbia ampio beneplacito, sia da parte dell'opposizione, sia da parte della stessa maggioranza. Quindi, stante l'assoluta importanza di pervenire a soluzioni concordate, auspico concreta e fattiva collaborazione fra tutte le forze politiche,

onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo Per le Autonomie approva e sostiene le linee guida del progetto di riforma che il Governo si accinge a presentare, illustrateci nell'intervento del ministro Mastella. Condividiamo i contenuti della sua relazione perché contiene l'indicazione di un progetto organico di riforma giudiziaria che abbraccia l'intervento sul processo e sull'ordinamento nel suo complesso. Come ho già sottolineato in quest'Aula della votazione sul provvedimento di parziale sospensione della riforma Castelli, questo Paese ha urgente necessità di una riforma che renda il sistema giustizia maggiormente garantista nei confronti dei diritti individuali e che rispetti il principio della divisione dei poteri e dell'indipendenza della magistratura. Il Paese ha, inoltre, palesemente bisogno di una riforma volta ad accelerare e semplificare i processi, perché la lentezza della nostra macchina giudiziaria è un problema serio al quale occorre trovare una soluzione tempestiva. Dobbiamo dunque garantire ai cittadini la possibilità di ottenere giustizia in tempi accettabili! Mi rincresce ripeterlo, ma nessuno dei provvedimenti varati dal precedente Governo mirava a rendere i processi più rapidi e la giustizia più efficiente per la generalità dei cittadini. L'Italia, infatti, occupa una delle posizioni peggiori nella classifica dell'efficienza del sistema giudiziario. Porre l'efficienza di tale sistema in cima alle proprie priorità non è soltanto necessario ma doveroso. Ringrazio, pertanto, il Ministro che intende ora rimediare a queste gravi mancanze e si accinge a varare provvedimenti volti all'accelerazione e alla semplificazione dei processi penali e civili, e misure di razionalizzazione della macchina giudiziaria a correggere norme *ad personam*, ossia norme forti con i deboli e supine con i forti. Come ha giustamente ricordato il ministro Mastella, il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Napolitano è inequivocabile e il Ministro ha ragione quando sostiene che la crisi di fiducia tra i cittadini e la giustizia è un problema causato anche dal confronto politico, troppo spesso acceso e strumentale. In materia di giustizia, trattandosi dell'effettività dei princìpi costituzionali di uguaglianza, di parità di fronte alla legge e di equilibrio dei poteri, è necessario uno sforzo di condivisione dei princìpi e smetterla con attacchi diretti ed indiretti alla libertà e all'autonomia della magistratura. Pertanto, esprimo, fin da subito l'augurio che il progetto di riforma, che il Governo presenterà e trasmetterà al Parlamento, possa diventare oggetto di una discussione seria e pacata tra maggioranza e opposizione. L'augurio, che esprimo, insomma, è che il confronto politico che si terrà in Parlamento dia un risultato ampiamente condiviso. Ciò servirà anche a ripristinare il rapporto di fiducia tra i cittadini ed il sistema giustizia. Riassumendo: l'obiettivo del progetto dovrà essere ridare efficienza al sistema giustizia e garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, così come prevede la Costituzione. Per concludere, signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie esprime la fiducia al Ministro della giustizia e approva la sua relazione e al tempo stesso la proposta di risoluzione presentata dalla senatrice Finocchiaro e dagli altri Capigruppo, noi inclusi,

sulla quale non si può che esprimere una valutazione positiva, impongono al Parlamento, in fase di riapertura dell'attività legislativa del 2007 e alla vigilia dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario, una riflessione sulle misure da adottare per riportare urgentemente l'effettività del servizio pubblico giustizia ad un livello elevato degno di una democrazia moderna e solidale, nel pieno rispetto della Costituzione. È dunque un bene che l'attenzione venga posta sul fatto che tutti i riti vigenti nel settore civile come nel penale non assicurino la ragionevole durata del processo prescritta dalla Costituzione e che finalmente si noti anche come, ad esempio, la Corte di cassazione rischi di affondare sotto il peso dell'arretrato giudiziario; ma il salto di qualità che ci attendiamo e che dobbiamo garantire ai cittadini va ben oltre le pur necessarie misure di riorganizzazione. Ad esempio, è vero che in molti dei distretti del Sud va rivista la distribuzione delle risorse e dei ruoli, ma una risposta alla criminalità organizzata non può esaurirsi nel contrasto di polizia, o peggio dell'Esercito, senza incidere sulle ragioni del radicamento economico, amministrativo e sociale dei fenomeni. Allo stesso modo, il provvedimento d'indulto, approvato a grande maggioranza dal Parlamento, deve essere necessariamente collocato in un più ampio contesto di iniziative finalizzate a ricondurre la pena nel dettato costituzionale. L'indulto, quindi, non può venir letto separatamente da un insieme di riforme da attuare a diverso livello ma tutte urgenti, poiché il settore giustizia non può essere visto come un qualsiasi ramo d'azienda in cui far quadrare i numeri e i bilanci separatamente dal contesto economico e sociale del Paese. Fa quindi bene la relazione del Ministro a sottolineare il mantenimento stabile del livello della popolazione detenuta a mesi ormai dal prodursi degli effetti dell'indulto; ma questo dato, che è doveroso ricordare, non può tranquillizzare nessuno: non è mantenendo stabile il numero dei detenuti che si misura la sicurezza sociale e la democrazia di un Paese. Per questo occorre procedere al rilancio di un nuovo modello di trattamento e detenzione sociale: dalle misure per le detenute madri alla sanità penitenziaria, misure che sono indispensabili per ristabilire da subito le condizioni minime di legalità nella fase di esecuzione della pena. Appoggiamo le prime iniziative assunte nel settore del lavoro e della sanità in ambito penitenziario, ma molti passi ancora debbono essere compiuti per rafforzare i diritti dei detenuti, a cominciare da una più ragionevole ed umana organizzazione dei trasferimenti. Anche in questo campo, oltre alle iniziative che il Governo vorrà mettere in campo, l'attenzione del Ministro della giustizia potrebbe utilmente rivolgersi al contenuto di numerose proposte di iniziativa particolare; ad esempio, le pene alternative, che sembrano assolutamente meritevoli di essere portati all'ordine del giorno dell'agenda politica. La situazione delle carceri italiane ha imposto un atto di clemenza, il quale ha avuto effetti - non dimentichiamolo - anzitutto su persone che stavano in carcere a causa di una dissennata politica repressiva, ma a questo punto occorre agire rapidamente e, in una certa misura modificare radicalmente, anzi, per rimuovere quelle norme che creano criminalità, anziché ridurla. La mancata contestuale dell'approvazione dell'amnistia, che ha avuto l'effetto paradossale di bloccare le aule processuali su processi ormai inutili - come hanno rilevato anche coloro che si sono opposti all'indulto e le diverse associazioni della magistratura e dell'avvocatura - dovrebbe indurci ad agire ancor più rapidamente per mettere mano a queste leggi. I tempi della giustizia siano dunque centrali nell'azione di Governo, ma i segnali che la politica deve rivolgere al Paese devono andare oltre. Si pensi ai familiari delle vittime delle stragi, ed in particolare al caso Ustica, che recentemente ha avuto una triste conclusione proprio sul piano processuale. È difficile negare che a quella brutta conclusione, alla quale si era cercato di dare un contributo, peggiorando, alla fine della scorsa legislatura, le norme penali che qualificano l'attentato contro gli organi costituzionali, di cui al comma 289 del codice penale, non si sia arrivati anche per l'inadeguata collaborazione delle istituzioni. Un segnale ora le istituzioni dovranno dare ai cittadini a distanza di quasi ventisette anni da quel 27 giugno 1980. Altre osservazioni per integrare l'analisi del Ministro: le norme riguardanti la giustizia in campo ambientale richiedono una rapida inversione di tendenza. Si pensi solo alle dissennate disposizioni sul danno ambientale e sulle bonifiche dei siti inquinati, alle norme premiali per l'abusivismo e alle ripetute ipotesi di depenalizzazione degli illeciti ambientali cui abbiamo dovuto assistere nella scorsa legislatura per comprendere quanto la centralità di questi temi debba essere recuperata. Il *business* dell'ecomafia dal 1994 ad oggi ammonta a quasi 180 miliardi di euro e i *clan* criminali coinvolti nell'illegalità ambientale sono oltre 200. Riteniamo quindi che nell'agenda delle iniziative legislative da approvare debba rientrare l'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale, facendo ciò che Paesi come Spagna e Germania hanno già fatto da tempo. Si tratterebbe di un'operazione di rilevanza epocale e dimostrerebbe un'inversione di tendenza in una legislazione improntata prevalentemente alla difesa degli interessi della produzione e quasi mai alle esigenze di tutela dell'ambiente. La dottrina più moderna e avanzata ha infatti notato come l'uso recente del termine «legge *ad personam*» ben si adatterebbe a norme che, da decenni, favoriscono specifici interessi o settori a scapito dell'ambiente, contando peraltro sulla debole natura contravvenzionale della quasi totalità dei reati ambientali, che costituisce una garanzia di impunità a causa dei tempi processuali. Alcune delle misure contenute nella legge finanziaria vanno in direzione del rafforzamento del sistema giustizia. Tuttavia, accanto agli interventi per snellire i tempi della giurisdizione, occorre fare attenzione a che talune misure non intervengano a scoraggiare il ricorso alla giustizia da parte dei cittadini, aggravando il costo degli strumenti processuali. Per questo non abbiamo valutato positivamente (c'era infatti anche un nostro emendamento che andava in senso diametralmente opposto) la disposizione contenuta nella legge finanziaria che ha aumentato il costo del contributo unificato per i ricorsi ai tribunali amministrativi e riteniamo che essa debba essere corretta, per evitare di far diventare il ricorso alla giustizia amministrativa, in particolare nel caso siano in gioco opere pubbliche o di pubbliche utilità, un rimedio dai costi insostenibili, soprattutto laddove si facciano valere interessi diffusi. Nel campo del processo del lavoro, le modifiche legislative intervenute nella precedente legislatura sugli istituti che regolano il rapporto di lavoro, in una fase di sua radicale trasformazione che vede il rapporto di lavoro subordinato diventare solo una delle varie possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa (in cui quello atipico viene assunto a modello contrattuale «normale»), hanno determinato riflessi negativi in relazione alla tutela dei diritti. Se appare grave la questione di diritto sostanziale, non meno preoccupante appare la situazione sotto il profilo processuale, dove si assiste, da un lato, alla tendenziale privatizzazione della giustizia del lavoro, dall'altro al tendenziale riassorbimento del rito del lavoro nel processo civile. I costi dell'arbitrato possono finire col rappresentare un disincentivo per i lavoratori a ricorrere alla giustizia. In sostanza, il problema principale della giustizia del lavoro è oggi, paradossalmente, che una gran parte di coloro che lavorano non ne ha accesso. In tal senso è positivo che, seppur timidamente, si sia cominciato ad attribuire a questi lavoratori garanzie e diritti da far valere anche in sede giurisdizionale, ricordando l'articolo 35 della Costituzione, per il quale «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». Per concludere, servono provvedimenti deflativi che blocchino la crescita del contenzioso arretrato e dei cosiddetti «tempi di giacenza», che giustamente la relazione del ministro definisce «indegni di un Paese civile». Ed è anche tempo di riflettere sull'andamento negativo dei tempi di dibattimento presso il giudice di pace, avendo ben chiaro però che ogni misura di semplificazione ed accelerazione dei processi deve essere compatibile con il mantenimento (anzi, il miglioramento) del livello qualitativo e quantitativo della tutela giurisdizionale dei diritti.

dare la nostra approvazione alla relazione del Ministro perché, come ho dimostrato, è assolutamente lacunosa, visto che egli si è limitato a prendere in esame soltanto alcuni aspetti di tutta l'attività

Ho assistito ad un dibattito paradossale, perché da tutte le parti si è levato un alto

dal 1996, riduce in termini assoluti e percentuali le risorse destinate alla giustizia in rapporto al bilancio dello Stato; allora, credo che un minimo di coerenza sarebbe necessaria. Guardiamo i fatti:

taglia pesantemente le risorse alla giustizia e castiga i professionisti. Il risultato è che i giudici di pace restano senza stipendio fatto mai accaduto durante il precedente Governo, noi abbiamo sempre pagato i magistrati, non abbiamo mai punito i professionisti. Il risultato è che i giudici di pace hanno fatto sciopero,

è aumentato fino ad arrivare all'1,7 del bilancio dello Stato. Per la prima volta quest'anno diminuisce, lo ripeto, in termini assoluti e percentuali. Pertanto, ritengo che una maggioranza che attua tali misure, evidentemente, non ami la giustizia.

Quindi, l'avete fatta nascere morta. Avete messo a capo di tale Commissione un parlamentare di prima nomina: il Presidente è totalmente inesperto dei meccanismi del Parlamento;

Se questo modo di andare avanti non cambia sostanzialmente, perché è ancora quello a cui ci hanno abituati in questi anni, se esso ha dimostrato che non ci porta fuori dalle secche di una giustizia lenta, perché accoglierlo? È evidente che non ci porterà da nessuna parte. Le segnalo un punto preciso su cui riflettere: mi riferisco alla questione del più stringente controllo sulla produttività dei magistrati, con la possibilità di espellere dalla classe dei magistrati coloro che vengono giudicati non all'altezza. Guardi che è esattamente il contrario del principio della libertà e dell'autonomia del magistrato, perché vuol dire renderlo schiavo in tutto e per tutto del CSM, cioè delle correnti, cioè dell'Associazione nazionale magistrati. Se passerà questo principio i magistrati saranno completamente succubi ai voleri delle correnti. Quindi, la invito veramente a meditare su questo punto; comunque avremo modo di discuterne quando il provvedimento verrà verrà in Parlamento. Chiudo con un'ultima questione. Lei ha fatto tanti voli pindarici, ma la invito ad utilizzare quello che già c'è, vale a dire le riforme che sono state fatte e votate anche in quest'Aula. Mi riferisco ai decreti legislativi di applicazione della riforma sull'ordinamento giudiziario: sono stati votati qui, mettiamoli in atto, usiamoli. Lei ha parlato tanto di efficienza

nell'intervento nella più alta sede, cioè l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di cassazione dell'anno scorso. Riferendosi alla possibilità di valutare gli uffici giudiziari e i magistrati, egli ha dichiarato: «In questo settore devo ricordare che si è avviato un proficuo lavoro tra il Consiglio superiore ed il Ministero della giustizia per elaborare efficaci criteri di controllo della produttività e della qualità del lavoro del magistrato, tenendo conto della pluralità delle funzioni. Questa esperienza di lavoro comune sembra essersi arenata, mentre meriterebbe certamente di essere sostenuta e potenziata». Signor Ministro, per aver varato questo progetto io mi sono preso una accusa di abuso d'ufficio, perché è vietato toccare il manovratore evidentemente; vedremo come andrà a finire, ma credo che questi rischi chi vuole fare politica credendoci e credendo nel proprio mandato, nella propria missione e nella missione del Parlamento li debba affrontare. Però l'arma in mano efficace lei ce l'ha: quindi, basta andare a vedere all'interno del Ministero quali sono già adesso le possibilità di andare avanti, senza bisogno di voli pindarici, senza bisogno dei sogni dei cinque anni. Lei ha

aveva la consapevolezza di essere assolutamente inferiore per quanto riguardava l'arma navale e allora radunò i generali e disse loro: ho trovato la soluzione; prosciughiamo la Manica, mandiamo la nostra Guardia imperiale, Cambronne, di là e invadiamo l'Inghilterra, perché siamo fortissimi con l'esercito di terra. I generali chiesero: ma come facciamo a prosciugare la Manica? E la risposta fu: dei particolari ve ne occupate voi, io elaboro le strategie. Ecco, non vorrei

L'aspetto della lunghezza del procedimento penale che ha portato all'assoluzione del collega Forte era una parte significativa, ma non era la parte politica del discorso. La parte politica del discorso era: perché è stato catturato nel 1993? La parte politica era: cosa è successo nel 1993? Su questo non c'è stata risposta, signor Ministro. Per questo non possiamo approvare la sua relazione: il silenzio su un punto per noi centrale della vicenda giudiziaria del nostro Paese ci inquieta molto e ci induce ad essere preoccupati sul futuro giudiziario di questo Paese. Quindi, non possiamo approvare la sua relazione per il silenzio che ha voluto mantenere nei confronti della domanda che ho posto. Chiedo ai colleghi dell'UDC di votare a favore

perché riguardano singole parti dell'ordinamento giudiziario sulle quali non abbiamo remore di nessun tipo. Abbiamo cercato di dare un contributo in questo ramo del Parlamento (come credo i colleghi del centro-sinistra possono ricordare, sia quelli della Commissione giustizia sia gli altri) quando si è trattato di discutere i disegni di legge relativi ai decreti legislativi sulle procure della Repubblica o sull'ordinamento disciplinare dei magistrati; abbiamo concorso a fare in modo che rimanessero in vita, modificati opportunamente. Altrettanto mi auguro che possiamo fare sull'ordinamento giudiziario: non abbiamo remore di contenuti a cercare un'intesa larga, ma siamo rammaricati del fatto che questa premessa in quest'Aula continui a non essere affrontata. Non ci si illuda. I problemi non risolti riemergono sia che si tratti del partito democratico che di quello unitario del centro-destra, sia che si tratti della natura e della idealità. Non ci si illuda che si possano ignorare i problemi politici non risolti. Mi auguro che da questo punto di vista il Ministro, al di là della sua personale simpatia, possa avere la forza di imporre alla sua maggioranza

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, in questa seconda parte del mio intervento, nel preannunciare il voto

accolte in questo suo programma, quando poi sarà esplicitato con atti legislativi. Innanzitutto, noi vorremmo, come detto anche da altri, che le carceri non tornassero a riempirsi in un breve periodo. Per ottenere ciò, bisognerebbe affrontare con grande determinazione il problema della depenalizzazione

Bossi-Fini sull'immigrazione, la ex Cirielli per la recidiva, la legge Fini-Giovanardi sulle droghe

Ritengo che qualsiasi riforma, qualsiasi speditezza di procedimento, qualsiasi aumento di garanzia giovi solo a chi può permettersi una difesa. Chi, invece, non può permettersi una difesa viene sempre stritolato cosicché l'efficienza della giustizia si risolve in assoluzioni o prescrizioni per chi ha una buona difesa e in una pena scontata interamente per chi non può avvalersi di una difesa degna di questo nome. Quindi, bisogna rivedere i veri meccanismi dell'accesso alla difesa con una vera riforma del gratuito patrocinio. Abbiamo anche noi il problema della Cassazione: riprenda il suo ruolo di stretta legittimità.

Quanto, poi, alla distribuzione dei tribunali, sono d'accordo sul fatto che la nostra mappa giudiziaria quella dell'Italia contadina, di cento anni fa. Se, però, lei si permette di spostare un solo tribunale, quell'Italia, con gli strumenti contadini del forcone e della falce, scenderà sotto il suo balcone al Ministero di via Arenula per protestare trasversalmente; trasversalmente; gli stessi elettori dell'onorevole Buccico saranno i primi a scendere in piazza, perché i tribunali non si toccano.

negazionismo, non abbiamo la coda di paglia, quindi siamo contro la penalizzazione di un reato di opinione. La *Shoah* è stato un episodio terribile della storia, che non ha bisogno di prove: queste sono costituite da quei milioni e milioni di cittadini che non abbiamo più incontrato dopo la fine della guerra

Lei presenta un programma che intende realizzare lo Stato di diritto e poi non ci dice niente su un procedimento penale

per cittadini americani che si sono macchiati di un grave delitto (il sequestro di persona) nel territorio italiano, senza bisogno di ricorso ai pentiti o ai servizi segreti, ma basandosi proprio sul lavoro della Polizia giudiziaria. giudiziaria. Respingere questa richiesta della magistratura di Milano sarebbe porsi sulla scia e nella cultura del passato Governo di centro-destra. Anche in questo campo non abbiamo nessuna coda di paglia: siamo contro il terrorismo e la violenza; abbiamo anche pagato in termini politici questa netta affermazione di contrarietà a qualsiasi tipo di violenza. quindi, che l'episodio di Abu Omar debba essere risolto all'interno dello regole di uno Stato di diritto

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il nostro passato, il passato della nostra cultura ha avuto radicamento su molte arti e tra queste su quelle dell'oratoria. I tempi nostri ci indicano che la questione è oggetto di un serio ripensamento e dunque la stringatezza dei discorsi è oggi considerata ragione di pregio degli stessi. Si parla sempre più spesso, anche nelle nostre istituzioni, di tempi europei; in questa logica, la risoluzione presentata dalla presidente senatrice Finocchiaro e dai Presidenti degli altri Gruppi dell'Unione sarebbe dunque da intendersi esemplare, tanto essa è stringata, definitiva, quasi sarebbe da dire icastica. Ma non è così. La risoluzione che la sua maggioranza le propone, signor Ministro, è figlia, esemplare rappresentazione dell'imbarazzo che le sue cosiddette comunicazioni determinano per chi abbia seria consapevolezza di quanto accade o di quanto non accade nelle giornate quotidiane nel mondo della nostra giustizia. Lei, signor Ministro, ha rimandato a futura memoria la reale rappresentazione al Parlamento di quanto realmente, quotidianamente accade o non accade negli uffici giudiziari del Paese, riparandosi dietro l'elenco delle poche cose fatte e proposte e dietro il nutrito elenco delle cose da fare, alcune davvero molto bizzarre, e ci conforta in proposito solo il fatto che lei è circondato, tra gli altri, anche da consiglieri fiduciari valenti, in cui riponiamo le nostre speranze perché lei non procuri più danni di quanti questo nostro Paese possa sopportare. Le cose che lei ha fatto: alcune le ha già ricordate nel proprio intervento il senatore Castelli, il quale è tornato su argomenti che più volte proposi, in più occasioni. Lei, signor Ministro, ha cinicamente liquidato, senza ragione e senza sua colpa, una sua Sottosegretaria che ebbe il torto, in materia d'indulto, di venire in Commissione giustizia e di leggere alcuni dati sul numero dei delinquenti da lei anzitempo restituiti ai cittadini (vi è anche da dire che lei, poi, recentemente, ha fatto scoppiare la pace con la Sottosegretaria stessa); lei, signor Ministro, si è invece tenuto stretto il sottosegretario Manconi, che ha evidentemente sposato come suo complice nel mentire al Parlamento, così come, ancora una volta lo ripeto, si è fatto più volte, anche con toni beffardi. Ci siamo opposti all'indulto conoscendo benissimo le situazioni di sovraffollamento nelle nostre carceri, abbiamo proposto che tra le varie soluzioni fosse quantomeno studiata e valutata quella - per così dire banale, banalissima - della commutazione di una parte della residua pena in detenzione domiciliare e non già della liberazione pura e semplice di chi era detenuto. Non se ne é neppure potuto parlare, perché evidentemente a lei e al suo sottosegretario Manconi altro interessava dal punto di vista politico. A Sollicciano, presidente Salvi, i nuovi detenuti post-indulto non sono affatto i soliti immigrati, cosiddette vittime della cosiddetta legge Bossi-Fini, ma sono, molto semplicemente, spacciatori che non hanno mai smesso di spacciare e seminare morte fra i nostri giovani e fra i nostri cittadini. Non prendiamoci in giro su argomenti come questi: sono argomenti su cui non c'è da scherzare. Le altre cose fatte, signor Ministro. Lei si è piegato sulle ragioni, si fa per dire (ed anche qui devo riprendere un tema già da altri proposto), del suo collega Bersani e non solo si è fatto espropriare di competenze mai prima d'ora poste in discussione

che non possano più essere pagati regolarmente quei giudici di pace che lei ora ci indica come soluzione ai problemi della giustizia, proponendo l'aumento della loro competenza e senza considerare che gli stessi lamentano, invece, l'aumento del rosso Provveda, signor Ministro, e in fretta, anche senza nessuna risoluzione sul punto. Non intendo ripetere oltre quanto molti altri colleghi hanno detto e quanto da noi scritto nelle proposte di risoluzione presentate dai colleghi Buccico, Valentino e dal ma quel che è certo è che Alleanza Nazionale non voterà la risoluzione proposta dalla sua maggioranza, che non ha nemmeno il coraggio di darle ragione. Si limita, infatti, a prendere atto e a non darle torto, come si usa forse fare in quella politica che non ci appartiene,

La prima è di procedere alla votazione con sistema elettronico sulla proposta di risoluzione n. 5, di cui mi permetto di leggere le poche righe del dispositivo per la ragione che è insita in ciò: «impegna il Governo, a proporre al Parlamento un disegno di legge di modifica costituzionale, che indichi, quale futuro assetto di sistema, quello della separazione delle carriere tra i giudici e i componenti dell'ufficio del pubblico ministero, con previsione di tutte le misure accessorie a tali scelte, perché possa essere avviato il dovuto dibattito parlamentare sulla questione; questione; a conferire puntuali indicazioni in tale direzione a tutti gli organismi italiani che operano in sede europea perché sia lì chiaramente indicato l'orientamento italiano sul tema».

a riprova di quanto ho testé affermato circa la volontà non ostruzionistica, avverto che se il numero legale dovesse mancare non insisteremo nella richiesta. Inoltre, signor Presidente, le chiedodi voler autorizzare la votazione per parti separate

di dover sottolineare che questo dibattito avrebbe avuto uno sviluppo molto più complesso, approfondito e consonante al dettato della legge se il Parlamento avesse avuto per tempo, non dico ventiquattro o dodici ore prima ma almeno qualche ora prima, non solo la relazione del Ministro ma soprattutto i dati afferenti all'attività dei Dipartimenti. Se si deve parlare dell'attuale stato della giustizia e del sistema giudiziario bisogna evidentemente conoscere questi dati. Tutto ciò non è stato possibile e la relazione del Ministro non si riferisce tanto al presente quanto al futuro, per cui, se del presente non si può parlare per mancanza di dati e per non avventurarsi in affermazioni prive di fondamento, parliamo del futuro.

che fino ad oggi hanno avuto scarso seguito. Al di là della legge di sospensione di alcuni decreti delegati della riforma Castelli,

crediamo alla sua buona volontà; l'abbiamo apprezzata e sperimentata positivamente nel confronto proficuo e costruttivo verificatosi in tema di ordinamento giudiziario in quest'Aula, ma a questo punto bisogna andare al concreto. Non è più

dei tempi di durata del processo. È necessario piuttosto confrontarsi sul concreto. Sul concreto consideriamo come sull'ordinamento giudiziario alla fine si scopre che i due decreti delegati, che non sono stati sospesi, sono a grandi linee quasi integralmente quelli varati dal ministro Castelli. Apprendiamo dalle sue dichiarazioni che a grandi linee la riforma a cui lei pensa ricalca il primo testo varato dal Senato sulla riforma dell'ordinamento giudiziario in ordine alla distinzione delle funzioni, alla qualificazione dei giudici, ai controlli e a tutto il resto, che fu aspramente combattuto dal centro-sinistra dell'epoca. Lei parla giustamente di maggiori controlli, di vigilanza, di qualificazione dei magistrati. Anche noi ne abbiamo parlato e chi non parlerebbe! Però non ha accettato il venir meno del condizionamento delle correnti sul CSM, il momento centrale di controllo dell'attività dei magistrati,

E oggi, malgrado prima il decreto Bersani e poi la finanziaria abbiamo apportato notevoli tagli al bilancio dell'amministrazione della giustizia con un risultato che rispetto alle precedenti occasioni è inferiore, nessuno protesta! Miracoli!

monumenti al sapere giuridico, ma che poi hanno scarsa capacità di raggiungere il concreto, visto che arrivano dopo anni e anni di tempo. di tempo. Dobbiamo poi andare avanti sulla informatizzazione certamente! Dobbiamo pensare anche ad una magistratura onoraria sempre più oberata che continua ad essere anch'essa molto precaria. Dobbiamo pensare ad una magistratura onoraria, in particolare ai giudici di pace sulla falsariga di quelli che erano i giudici conciliatori o oggi giudici tributari, che durano in carica, salvo revoca, assicurando anche quella esperienza e quella possibilità di continuità giurisprudenziale indispensabile ed evitando esperienze nuove. Sul processo penale abbiamo sentito poche considerazioni interessanti, ma non abbiamo capito il sistema nuovo, se vi sarà: estrema genericità! Sulla giustizia minorile dobbiamo uscire dall'equivoco: se non si investe nel sistema del rapporto tra famiglia e minore che delinque, non possiamo uscirne e dovremo fare ricorso ad una maggiore severità.

Nulla sulle politiche penitenziarie: il problema è quello di realizzare rapidamente nuove carceri, ma soprattutto di investire sulla rieducazione, sul reinserimento, sulla capacità di assicurare dignità, sicurezza e ovviamente assistenza sanitaria all'interno delle carceri. Sui professionisti, signor Ministro, se è vero è riuscito a varare una riforma complessiva delle professioni rimane però quella asportazione fatta con destrezza politica dal suo collega Bersani che tanti problemi ha creato ai professionisti nel lodevole intento di combattere l'evasione fiscale, creando una farraginosità di rapporti con i clienti che alla fine non credo gioveranno molto a questo tipo di lotta che tutti dobbiamo portare avanti. Ma andiamo al problema vero, al problema vero, quello finanziario, come sempre. Finché ci saranno tagli all'amministrazione della giustizia tutte queste riforme non potranno mai arrivare a compimento, non potranno mai essere attuate, perché le riforme di sistema, di sistema, di modifica del diritto sostanziale e anche del rito hanno necessità di funzionari amministrativi, di giudici qualificati, di mezzi e strumenti che oggi, purtroppo, sono carenti.

crisi e di bisogno dei vari uffici giudiziari e soprattutto non si parla del cosiddetto ufficio del giudice, che era utile a far venire meno una serie di attività per certi versi preparatorie ma alla fine defatiganti e che allungavano i tempi delle decisioni. Anche qui c'è necessità di investimenti e di far venire meno quel precariato che oggi regge concretamente tutti gli uffici giudiziari. I precari sono circa 1.800 in tutta Italia, 260 solo a Palermo; senza di loro questi uffici giudiziari Senza tali investimenti, senza la capacità di pesare nell'ambito del Governo, di porre al centro del programma il sistema giustizia, noi non ne usciremo.

Allo stato la nostra è una valutazione negativa e pertanto voteremo contro, ma siamo pronti a ricrederci. Siamo aperti al dialogo concreto e la attendiamo nella concretezza dei fatti. Lo abbiamo dimostrato, il dialogo costruttivo nell'interesse del Paese è nel nostro DNA. Nella nostra proposta di risoluzione non abbiamo chiesto la luna, tant'è che lei ha

rigorosamente ancorato alle competenze istituzionali del Ministro della giustizia, che, sulla base dell'articolo 110 della Costituzione, riguardano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Correttamente il Ministro non ha quindi fatto riferimento, né alle linee che emergono dalla giurisprudenza, sia nel campo penale e civile nell'anno che ora si conclude, né a una funzione di tipo giudiziario, che pure in qualche misura gli appartiene, quella di controllo disciplinare. Egli ci ha parlato soltanto dell'organizzazione del sistema giustizia e dei programmi e delle intenzioni che sono proprie del Ministro e del Governo in questo campo. Per quanto riguarda l'organizzazione, voglio sottolineare quanto significativi siano i dati che il Ministro ci ha fornito circa le risorse destinate negli ultimi anni alla giustizia. Qui davvero c'è bisogno di un ripensamento che deve essere comune a tutti noi e che deve indurci a mutare direzione, a cambiare atteggiamento, perché il sistema giustizia è stato sottoposto negli ultimi anni a un progressivo depauperamento dei fondi e delle risorse. Invece vi sono spese, come quelle relative al sistema giudiziario, che non possono essere compresse oltre un certo limite perché questa compressione determina uno scadimento nel livello di vita civile del Paese. Quando vedo che tra il 2005 e il 2006 vi è stata una diminuzione nelle risorse stanziate di 53 milioni di euro euro mi trovo di fronte a un fatto straordinario, a una svolta in senso regressivo. L'impegno del Governo di centro-sinistra nei prossimi anni deve essere volto a invertire tale tendenza. Certamente, nella finanziaria del 2007 vedo già un milione di euro in più rispetto ai dati della finanziaria dell'anno precedente, cioè dell'ultimo anno del Governo della passata legislatura. Questo, evidentemente, non basta:

voi sapete che nell'ambito di un procedimento penale istituito presso gli uffici giudiziari di Milano per un reato grave, il sequestro di persona, è stata avanzata la richiesta di estradizione di un numero piuttosto elevato di cittadini americani (oltre venti) appartenenti all'*intelligence* di quel Paese, indagati per sequestro di persona e nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare. Il sequestro di Abu Omar è un fatto grave, perché con quell'azione clandestina si è sottratto un sospetto di terrorismo alle indagini che nei suoi confronti si stavano svolgendo e che erano dirette dall'autorità giudiziaria giudiziaria competente. È un fatto grave perché la lotta contro il terrorismo non deve essere mai - a nostro giudizio - condotta calpestando i diritti fondamentali delle persone; altrimenti, ci mettiamo allo stesso livello dei il punto di vista europeo è quello ed è stato ribadito più volte: quel procedimento penale, signor Ministro, ha una certa importanza. Noi le chiediamo di decidere sulla richiesta di estradizione.

Spieghi al Parlamento e all'opinione pubblica le ragioni della sua decisione. Signor Ministro, con viva amicizia le diciamo: non c'è niente di peggio del silenzio. Bisogna decidere, nell'uno o nell'altro senso e poi, con franchezza (perché è sempre bene dire la verità) spiegare al Parlamento e all'opinione pubblica le ragioni della propria decisione. Alcune questioni sono state al centro delle proposte programmatiche che il Ministro ci ha sottoposto: in primo luogo, i tempi della giustizia. Noi chiediamo al Ministro e ai colleghi di lavorare insieme perché presto si possa istituire una vera e propria sessione parlamentare, un dibattito organico che riguardi più provvedimenti

La questione dei tempi della giustizia è centrale per l'opinione pubblica e per i cittadini: una giustizia che arriva tardi non è giustizia. Concentriamo tutti i nostri sforzi su tale priorità. Le proposte ci sono:

C'è bisogno di una semplificazione del processo civile, di tagliare i tempi morti del processo penale e di una nuova disciplina delle nullità. Ebbene, tutti questi provvedimenti, tutte queste proposte possano trovare un alveo comune in una sessione parlamentare e si comunichi al Paese che si ha intenzione di lavorare una settimana o dieci giorni per approntare una normativa nuova che punti da più lati ad accelerare i tempi della giustizia. giustizia. Proprio un'ora fa ci è giunta notizia, signor Presidente, che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la cosiddetta legge Pecorella, quella che stabiliva la inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero. I motivi per i quali questa legge viene dichiarata incostituzionale, per quel che possiamo comprendere dal dispositivo - ma senz'altro leggeremo il testo della sentenza -, sono gli stessi che noi

riteneva di poter interpretare e che i suoi sostenitori hanno sbandierato. In verità, essa è in contrasto con il principio di parità delle parti nel processo e non è tale da tutelare i diritti delle parti lese. Leggeremo, comunque, quella sentenza e vedremo se da essa scaturiscono indicazioni utili per il legislatore, per tornare sopra queste disposizioni che la Corte costituzionale ha messo nel nulla. Per quel che riguarda il processo penale, vi sono altre leggi che sono state fonte di allungamento dei tempi e di ingiustizia.

dallo scontro preconcetto, al fine di intervenire su norme che sono, evidentemente, irragionevoli e che richiedono necessariamente una modificazione, in qualche caso una modificazione profonda. Le norme in materia di prescrizione, contenute nella cosiddetta legge ex Cirielli, sono irragionevoli e prescindono dalle esigenze particolari che allora le dettarono. Il fatto è che queste norme non possono rimanere nell'ordinamento italiano perché sono fonte di disordine. Ho apprezzato le proposte del Ministro della giustizia in tema di ordinamento giudiziario, così come ho trovato interessante così come ho trovato interessante e condivisibile la parte della sua relazione che si riferisce alla giustizia minorile. Voglio però dirle, signor Ministro, che è tempo di passare al concreto lavoro legislativo. Le proposte ci sono, la linea che emerge dalla sua relazione è limpida e, ascoltando il dibattito (a parte le ovvie prese di posizione politiche), ho l'impressione che si possa costruire, sulla linea da lei enunciata, un consenso ampio, una discussione serena, che si possa giungere in molti casi a conclusioni condivise. Dunque, al lavoro; al lavoro in Parlamento sulla base delle proposte che il Governo ci ha qui illustrato.

con l'intesa che l'esito di ciascuno dei voti non sarà ostativo alla votazione delle risoluzioni successive che si intenderanno messe ai voti per le parti, eventualmente, non precluse, né assorbite.

Io mi inchino alle osservazioni del senatore Boccia, che evidentemente sono più puntuali di quanto non sia stato da noi scritto. Volevo solo precisare all'Assemblea e al signor Ministro che intendevamo dire la legge finanziaria che sarà votata nel 2007 e che quindi si riferirà all'esercizio 2008.

all'apertura della seduta pomeridiana, il Senato ha approvato a larga maggioranza le due mozioni riguardanti la Libia, con il parere del Governo favorevole per entrambe. A una

nell'ultimo capoverso del dispositivo che impegna il Governo. Quel paragrafo, così come approvato alle ore 16, «impegna il Governo a risolvere in tempi ragionevoli le questioni relative ai crediti dei cittadini italiani per i beni impegnati in attività libiche». Al fine di poter operare, il Ministero degli affari esteri ha chiesto - e concordiamo - che quelle due righe si leggano nel modo seguente: «a risolvere in tempi ragionevoli le problematiche concernenti i profughi italiani in Libia e le questioni relative ai crediti delle società italiane nei confronti di Amministrazioni ed Enti libici». Su tale linguaggio credo vi sia

Presidente Dini, il dispositivo è quello che è stato votato, ma trattandosi di una mozione, e dunque di un impegno al Governo, sarà

Signor Presidente, sento il dovere di comunicare all'Aula un fatto gravissimo accaduto poche ore fa in Calabria. Si è tenuta a Catanzaro una manifestazione di lavoratori precari e sono avvenuti degli scontri: purtroppo, vi è stato un attacco durissimo e particolarmente violento da parte delle forze dell'ordine contro i lavoratori, manganellate in testa, teste rotte e diversi feriti, alcuni dei quali finiti in ospedale. A nome del Gruppo di Rifondazione Comunista sento di dover stigmatizzare severamente questo operato.